siamo qui oggi per compiere l'ultimo atto parlamentare, il passaggio definitivo, per l'approvazione del disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011» (sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012), già approvato dalla Camera dei deputati il 28 maggio scorso.

per la convinzione con la quale hanno voluto esprimere un voto unanime, così come i colleghi di tutte le altre Commissioni che hanno espresso pareri favorevoli. La ratifica di questa Convenzione rappresenta un atto di grande importanza. Esso è il risultato dell'intenso lavoro delle parlamentari italiane: quelle che hanno operato all'interno del Consiglio d'Europa perché si arrivasse alla Convenzione, quelle che, con il loro lavoro, quasi a conclusione della scorsa legislatura, sono riuscite ad avviare il dibattito qui in Senato ed a conquistare la firma del Governo italiano;

importante. Con la Convenzione siamo allora di fronte a uno strumento nuovo, più vicino ai fatti che alle parole, ai tanti appelli e alle tante risoluzioni di condanna; uno strumento che, una volta operativo, sarà per la prima volta giuridicamente vincolante per un'efficace lotta alla violenza contro le donne in termini di prevenzione, protezione, repressione, monitoraggio e integrazione delle politiche; il primo e più avanzato strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.

ha visto leggi importanti, ottenute con il concorso, come dirò più avanti, di tutte le culture politiche, che sono una grande ricchezza e un valore molto importante della nostra tradizione giuridica. La Convenzione è il primo trattato che riconosce la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione, configurandola dunque come violazione del principio di uguaglianza. Questo è il nocciolo della Convenzione, su cui tornerò. È il riconoscimento implicito della necessità di mettere in campo qualsiasi strumento che incida profondamente sulla cultura, l'educazione, l'istruzione e la comunicazione e che intervenga, contestualmente, in tutti gli aspetti della vita che davvero possono determinare parità ed uguaglianza.

perché quando diventa coscienza comune non dobbiamo illuderci che il problema, non dico non esista più, ma neanche che non sia importante, come mi sembra di registrare dal brusìo. Personalmente, diffido sempre della facile indignazione e dell'unanimismo, perché il clamore dei *media*, il fatto di averne sentito parlare tante volte e l'unanime sdegno (chi è infatti

ottenendo l'effetto opposto fino ad arrivare addirittura a forme di negazionismo, come abbiamo visto anche recentemente, proprio come reazione ad un eccesso di

di non farne un oggetto di moda quanto poco veramente sentito, di non avere un atteggiamento vittimistico o vendicativo, perché se rimaniamo fermi e lucidi possiamo individuare le misure legislative adeguate, come sta già avvenendo con i nuovi decreti. Questa lucidità nel non esagerare nell'aspetto propagandistico

e che i dati quantitativi e qualitativi dei crimini confermano che si tratta di una vera e propria piaga sociale che riguarda donne di tutti i ceti sociali, di tutte le età ed è presente nelle società avanzate come in quelle arretrate. da tempo non riguarda casi estremi o platealmente efferati, ma che purtroppo nasce nel cuore stesso della relazione tra i sessi e nella stessa vita familiare. La Convenzione coglie molto bene questo aspetto di domesticità e di orrore domestico perché lo riconduce alla violenza in ambito domestico, che non colpisce per questa natura solo le donne, ma anche i bambini e gli anziani, ai quali si applicano infatti le medesime misure di tutela. A conferma di ciò, nel preambolo si sottolinea che il raggiungimento dell'uguaglianza tra i sessi *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne. Vorrei qui sottolineare i due punti qualificanti che sono la vera novità della Convenzione, che introducono davvero aspetti inediti e che sono presenti nel preambolo e nell'articolo 3, che è quello più ricco il primo punto riguarda il nesso tra diritti umani e violenza contro le donne e il fatto che essa sia causa e conseguenza dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi. i sessi. Lo spirito, la filosofia della Convenzione è allora quella di combattere la violenza contro le donne secondo il principio per il quale i diritti umani sono ormai il vero banco di prova del livello di civiltà dei nostri Paesi non meno che le questioni economiche o angustamente nazionali. Questo ci riporta alla natura e alla nuova qualità dei diritti umani oggi. Il secondo punto riguarda il tema della parità tra i sessi. gli sconfortanti dati della condizione sociale, culturale e lavorativa delle donne del nostro Paese dimostrano che molta strada abbiamo da fare su questo terreno.

Molti parlano di stereotipi e di pregiudizi, ma la questione è più profonda e sottile insieme. Non riguarda solo qualche comportamento arretrato, possessivo e violento, con cui prende forma la tradizionale gelosia maschile, almeno non nei nostri Paesi, non in Italia e non in Europa. L'efferatezza, ma anche l'ordinaria banalità di crimini mostruosi, come quelli perpetrati dagli adolescenti sulle loro coetanee o i normali compagni nella vita domestica sulle madri dei loro figli, tutto questo orrore rimanda alla natura della crisi culturale e morale che stiamo vivendo nella quale prosperano rapporti di forza disuguali.

su una donna divenuta troppo forte, che vuole scegliere autonomamente. Ed è su un altro aspetto che vorrei richiamare la vostra attenzione: cioè sul complicato nesso tra uguaglianza con l'uomo e differenza femminile, perché è in esso che si annidano le vere sfide, le vere insidie culturali e psicologiche, quelle più difficili da decifrare e quindi da sconfiggere, da debellare. Quando si dice, e giustamente, che non bastano le leggi per arginare il fenomeno della violenza contro le donne, perché occorrerebbe andare anche alle sue radici culturali, non si deve intendere secondo me allora solo e tanto i cosiddetti pregiudizi o stereotipi. Questa è una lettura di superficie. L'esplosione di queste variegate forme di violenza rimanda a una natura profonda della crisi di identità della soggettività maschile, ad una sorta di destabilizzazione dell'uomo verso quella strana e inedita identità femminile che lo spaventa, perché insieme alle richieste di uguaglianza la donna rivendica anche, sempre e ancora di più una sua specificità tutta femminile. Le donne vogliono la parità, certo, e quindi la libertà di decidere e di scegliere, senza rinunciare però alle loro prerogative specificatamente femminili. Una creatura strana, dunque, la donna di oggi: forte, molto forte eppure molto femminile. Tutto ciò disorienta e spaventa l'uomo, provocando una vera e propria crisi di relazione tra i sessi. Scusate questa parentesi, ma spesso non si colgono le radici profonde del fenomeno. donne sta la precondizione essenziale e necessaria per prevenire la violenza di genere. Ora mi sembra doveroso fare alcuni approfondimenti, anche se per una disamina approfondita del testo degli articoli della Convenzione rimando al testo scritto. rapidamente - si compone di un preambolo che raccoglie il senso di cui dicevo prima, il nesso con i diritti umani, e 81 articoli divisi in 12 capitoli. L'obiettivo della Convenzione, contenuto nell'articolo 1, che segue al preambolo, è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne, nonché la cooperazione internazionale (che è il quadro fondamentale in cui tutto ciò si coglie, per questo è importante che venga ratificato da

che come sappiamo è la circostanza in cui c'è una recrudescenza feroce della violenza. Lo sappiamo dalla storia recente e quella passata: il corpo femminile durante la guerra, con gli stupri, è metonimico, metaforico della violenza e del possesso dell'uomo sulla Patria che sulla Patria che deve difendere e sulla Patria che deve conquistare. Questo è stato vero nelle guerre mondiali, ma lo abbiamo visto anche nella guerra del Kosovo e nel *post* conflitto dopo l'eccidio in Ruanda. Dunque, è molto importante questo quadro, che infatti si riferisce a tutti i Paesi del mondo e a tutte le condizioni di pace e di guerra. L'articolo 3 contiene una serie di definizioni e di termini,

per fare riferimento - cito - a «ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini ». Ho riportato la citazione per intero perché questa definizione, come sapete, ha suscitato parecchie polemiche, che si sono poi unanimemente concluse con l'affermazione che «l'Italia applicherà la Convenzione in conformità con i principi della Costituzione italiana». Sorvolo su tanti capitoli e mi soffermo solo sul capitolo, si dilunga abbondantemente su una serie di impegni che riguardano il metodo con cui gli Stati si impegnano ad affrontare il fenomeno. In questo caso, tra l'altro, si fa riferimento ‑ ed è molto importante per noi ‑ all'esigenza di coordinamento delle diverse politiche e al coinvolgimento delle organizzazioni non governative della società civile, alla raccolta dei dati, alla prevenzione, e tutto quello che costituisce la ricchezza e il contenuto migliore della Convenzione. Tra questi temi, ampio spazio è dato alla prevenzione, cui è dedicato il terzo capitolo, anch'esso molto importante in La prevenzione richiederebbe una discussione a sé, che non faccio e che spero e penso sicuramente sarà ripresa nel corso Il cuore della prevenzione, infatti, com'è chiaro, non può essere propriamente giuridico. La prevenzione è un fatto - come ho già detto prima - culturale, morale, psicologico,

a questo tipo di reazioni incontrollate e inconsulte. Se quindi - come dicevamo - siamo di fronte a realtà complesse e profonde, ciò non toglie, ovviamente, che ci si debba impegnare - e la Convenzione lo fa molto bene - per adottare per adottare misure in senso preventivo, che siano legate alla campagna di sensibilizzazione (ne parla diffusamente l'articolo 13), a programmi educativi, al controllo sull'uso dell'immagine femminile del corpo, e via dicendo. Si tratta di temi che richiedono anche figure professionali preparate e formate *ad hoc*.

alle case rifugio, ai centri antiviolenza, alle linee telefoniche, tutto un apparato di protezione che ha nel volontariato le larghe basi, ma che non può essere abbandonato a sé stesso, e non solo sul piano dei

Un altro elemento interessante, che non era presente in alcuna Convenzione internazionale, è la specificazione della sede dei reati, tra cui rientra la violenza psicologica, l'aborto forzato, le molestie e il matrimonio forzato, che, come sapete, ha grandissima importanza in tantissimi Paesi La Convenzione chiede che gli Stati si impegnino a introdurre nei propri ordinamenti, qualora non ci fossero, per i quali devono essere predisposte sanzioni definite «efficaci, proporzionate e dissuasive», quindi non vendicative, ma molto più stringenti.

nel recente decreto del nostro Governo. Si tratta del capitolo VII dedicato alle donne migranti e alle donne richiedenti asilo: due categorie che, come potete ben capire, sono particolarmente soggette a violenze di genere.

di ottenere uno *status* di residente indipendente da quello del coniuge e del *partner*: questo è molto importante e - ripeto - è un passaggio che ha già trovato buon riscontro nei decreti emanati due giorni fa dal nostro Governo. Inoltre, viene stabilito l'obbligo di riconoscere la violenza di genere come una forma di persecuzione - ai sensi della Convenzione del 1951 sullo *status* dei rifugiati - e viene ribadito l'obbligo di rispettare il diritto al non respingimento per le vittime di violenza contro le donne.

Prima di concludere, mi preme chiarire fin da subito due punti. con un atto finale, che segue un processo di discussione non solo legislativa, è un tipo di strumento che ci richiede una ratifica «secca», cioè le norme di adeguamento dell'ordinamento interno. La scelta di questo strumento si giustifica con la volontà di pervenire nei tempi più rapidi possibili alla ratifica da parte del nostro Paese. Paese, ma questo non deve essere scambiato per una scelta rinunciataria. Questo non significa accontentarsi della ratifica - che è importante e la rapidità con cui la facciamo è strumentale ed è «secca» perché la vogliamo avere subito, velocemente - o che non dobbiamo occuparci degli impegni che la Convenzione richiede. Questa è la prima cosa di cui dobbiamo essere responsabili in questa scelta. Il secondo Il secondo punto, che è la conseguenza di questo, riguarda le risorse finanziarie. Non voglio riaprire la questione della copertura finanziaria, che è stata già affrontata dalla Commissione bilancio e discussa ampiamente alla Camera. Commissione ha subordinato il proprio parere favorevole all'inserimento della clausola di neutralità finanziaria, ora contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge.

In questo senso, penso, potrebbe essere molto utile la proposta della ministra Idem di una *task force* che potrebbe drenare nei vari Ministeri delle risorse. risorse. Voglio concludere dicendo che dobbiamo esprimere un pronunciamento unitario e convinto e non semplicemente un assenso, come si usa dire banalmente, *bipartisan* La nostra legislazione ha una tradizione prestigiosissima in tema di diritto di famiglia, di tutela delle donne e dei minori. Penso al diritto di famiglia, alla legge contro la violenza sulle donne e a quella anti *stalking*. Queste sono state il frutto delle migliori culture politiche del nostro Paese e non solo giuridiche. Di queste culture, oggi esaurite in parte o, comunque, esauste, dobbiamo recuperare il lascito migliore, senza nostalgie, ma neppure rimozioni demolitorie che ci consegnano il nulla. Seppur apprezziamo il testo della Convenzione, proprio per questa ricchezza ne vediamo anche gli aspetti forse troppo formali e in parte algidi che andrebbero innervati con lo spessore delle nostre convinzioni e della nostra tradizione italiana dove grande peso hanno e possono avere le relazioni buone tra i sessi, le generazioni e le famiglie. famiglie. Qual è la lezione migliore che possiamo trarre da questo innervamento tra la nostra tradizione e lo spirito europeo? Lo dico in tre punti. La nostra lezione La nostra lezione è fare sì che la sensibilità legislativa, nostra, italiana su questi temi, come sui diritti umani in generale, sia inversamente proporzionale alla scarsa o nulla applicazione pratica, concreta e reale di questi dettami nella vita concreta delle nostre donne. In secondo luogo, bisogna fare sì che essere il che essere il secondo Paese dell'Unione europea che ratifica la Convenzione ci impegni a debellare la nostra casistica che è tra le più allarmanti d'Europa sulla violenza di genere per numero di vittime ed efferatezza dei crimini. fare sì che la parità tra uomini e donne diventi reale e non solo enunciata e che questo non rappresenti un ennesimo piano di scontro, questa volta tra i sessi, ma una comune consapevolezza che veda gli uomini per primi impegnati contro questa odiosa violenza. Insomma, colleghe, colleghi, Presidente, ratifichiamo questa Convenzione non come uno stanco e rituale gesto politicamente corretto, ma con la convinzione, di cuore e di testa, che queste sono battaglie vere, per animare una civiltà esausta non solo a causa della crisi economica ma, anche, dal venir meno dei principi basilari di un comune umanesimo che non potrà mai più prescindere dal riconoscimento dei diritti di un pieno e libero umanesimo femminile. **Congedi e

Oggi intervengo in quest'Aula con un'apprensione particolare e una partecipazione vera, molto sentita. La questione che ora affrontiamo non è più eludibile e ha ormai assunto i contorni di una vera e propria emergenza sociale, culturale e, e, quindi, anche politica: la violenza nei confronti delle donne. In questa fase illustrerò dunque la mozione che ha presentato il Gruppo Lega Nord e Autonomie,

tocca un tema che ci vede tutti coinvolti, onorevoli colleghi, uomini e donne, in una battaglia comune che è soprattutto e prima di tutto una battaglia culturale rispetto alla quale la sensibilità del nostro Gruppo è caratterizzata da una particolare attenzione che vuole essere per questo che abbiamo voluto presentare subito, prontamente una mozione specifica che nel suo contenuto, molto articolato e suddiviso per

sul tema. La nostra mozione fa riferimento al tema della prevenzione, della protezione delle vittime ma anche e soprattutto ad un aspetto in questo momento particolarmente importante, quello delle sanzioni, della repressione e delle misure di carattere

regime sanzionatorio deve avere. Gli episodi tragici, brutali ai quali abbiamo assistito e assistiamo quotidianamente per la crudeltà e l'accanimento con cui vengono esercitati meritano di fatto, anche da un punto di vista giudiziario, penale e sanzionatorio,

pensando a forme di indulto e di amnistia che porterebbero fuori dalle carceri proprio coloro che si macchiano di questi reati infamanti. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, PdL e M5S)*. E voglio anche in questa occasione sottolineare la nostra massima attenzione. Non è infatti pensabile che introduciamo nell'ordinamento

non si riesce ad affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri. Nel nostro Paese, se da un lato negli ultimi dieci anni il numero complessivo degli omicidi è diminuito, lato va sottolineato che il numero degli omicidi perpetrati nei confronti delle donne è aumentato, ed è aumentato in maniera allarmante. I dati del 2012 indicano che in Italia si sono registrate più di 120 vittime. Nella maggior parte dei casi gli autori di tali delitti sono legati alle vittime da un rapporto familiare, ossia da un rapporto parentale: il più delle volte casi di questo tipo (violenze perpetrate dal punto di vista fisico e psicologico o soprusi nei confronti delle donne)

bene, quindi, arrivare alla ratifica della Convenzione di Istanbul, di cui parleremo dopo, che segna senz'altro un passo avanti davvero importante. Vorrei segnalare però che questa Convenzione

rende quindi necessaria l'introduzione nel codice penale di una fattispecie di reato *ad hoc*, che è appunto quella del reato di femminicidio. La circostanza che i delitti vengano perpetrati, per lo più, sulla base di una relazione di affetto o conoscenza di una donna esplicita una dimensione sociale della violenza che va veramente analizzata e ci porta ad affermare chiaramente che la repressione, la punizione in maniera efficace e rigorosa dei colpevoli non è certamente sufficiente. Occorre agire sul fronte della prevenzione e soprattutto su quello dell'educazione culturale, facendo fare finalmente

che richiamano la nostra attenzione su quello che deve essere un approccio diverso dal punto di vista culturale. Nel nostro Paese, nonostante l'entità drammaticamente allarmante del fenomeno, esempio - una commissione preposta all'analisi e al monitoraggio dei dati relativi alla violenza contro le donne. Si tratta di una lacuna che però si somma ad altre problematiche, rispetto alle quali con la nostra mozione intendiamo richiamare l'attenzione del Governo -

Se i fatti criminosi di violenza contro le donne (violenza fisica ma anche psicologica) avvengono in un contesto familiare domestico, bisogna ricordare che sono spesso legati anche a una situazione di impotenza delle donne dal punto di vista economico, di incapacità a mantenersi. anche investendo molto sulla formazione nelle scuole e negli istituti scolastici, ma anche sul fronte delle risorse, che devono essere assolutamente recuperate per dare sostegno ai centri antiviolenza e agli istituti di protezione, che sono assolutamente fondamentali perché sul territorio danno un contributo vero a tutte le donne vittime di violenza. Chiediamo quindi al Governo di impegnarsi a proseguire il programma diretto a contrastare il fenomeno della violenza donne promuovendo, anche attraverso appositi finanziamenti, il sostegno delle rette dei centri antiviolenza presenti sul territorio nazionale; a mettere in atto iniziative volte a promuovere la conoscenza e l'applicazione effettiva della normativa in tema di violenza di genere; più efficaci, dal punto di vista processuale e ordinamentale, per contrastare in modo concreto tutte queste forme di violenza contro le donne e ad assumere con celerità, anche nei processi, la visione di quanto sia indispensabile garantire un'efficace tutela giudiziaria alle vittime. Pertanto, con la mozione n. 56, che spero possa essere condivisa e sottoscritta da altri colleghi, chiediamo un impegno preciso al Governo perché non è più possibile considerare questo fenomeno semplicemente

io esprimo molta soddisfazione perché, in fondo, all'inizio di questa legislatura ci occupiamo di un tema così importante e delicato: è stato fatto alla Camera e lo facciamo al Senato.

La Convenzione contiene anche innovazioni che possono e dovranno stimolare il nostro ordinamento:

Noi abbiamo voluto inserire in un disegno di legge la circostanza aggravante di femminicidio, il cosiddetto reato di femminicidio, che non incide solo sull'omicidio ma viene spalmato su vari articoli del codice Ciò è importante per dare un segnale preciso in termini di violenza di genere, che non è solo violenza domestica. Vorrei altresì ricordare un dato molto importante, affinché non rimangano solo parole. È vero, come diceva la collega, il dato economico. Mi dispiace che non ci sia il Ministro delle pari opportunità

per questo universo, che è il reato contro le donne, la violenza contro le donne, ha un costo.

una sproporzione sia quantitativa che qualitativa tra accusa e difesa. Colleghi, è molto importante che sia ribadito questo principio. Tra l'altro, c'è un'innovazione, una riflessione della Convenzione molto importante, che richiamiamo anche nelle mozioni,

donne, e non solo, che si sono suicidate per contenuti degradanti all'interno di Internet. Ecco, anche su questo dobbiamo essere pronti con una legge che sia all'avanguardia, al passo con i tempi. Ripeto, fermo restando il diritto alla libera espressione, non ci deve essere violenza di contenuti formali contro donne e bambini, soprattutto per quanto riguarda la Rete, che è diventata un oggetto quasi del desiderio, un elemento importantissimo, uno strumento importante.

di violenza - non cominciamo a parlare, ad agire e a fare finalmente una legge contro la prostituzione, per regolamentare la prostituzione? Perché continuiamo a fare finta che che non esista e chiudiamo gli occhi, quando ognuno di noi nel proprio Comune vede questo fenomeno così grave, con ragazze sempre più piccole? Bisogna affrontarlo, e nelle scorse legislature eravamo quasi a un passo

del nostro ordinamento rispetto alla Convenzione di Istanbul. Questo si deve fare, e sollecito anche, come è stato rilevato, una struttura interministeriale, perché delle donne, così come dei bambini, non se ne occupa nessuno: nessun Ministero ha in realtà una competenza specifica, perché in fondo - se non gli hanno cambiato la delega - il Ministro delle pari opportunità ha una delega limitata alla prostituzione femminile. E inoltre, colleghi, io volevo qui sollecitarvi su un punto, lo devo dire. Ricordiamoci che noi siamo all'avanguardia rispetto a molte leggi, anche in Europa. Io non voglio usare un termine, ma voglio richiamare l'attenzione su un punto. Se avete il testo della Convenzione, colleghe e colleghi, andate a vedere all'articolo 36

come e quando, perché una donna, durante il processo, non deve di nuovo subire un interrogatorio morboso e perverso, se c'è una cosa o meno. E non lo voglio dire che cosa c'è. E invece purtroppo nella Convenzione si ritorna a questo concetto antico; lo dovete andare a vedere. Io sono rimasta un pochino, non dico perplessa, ma molto di più. Attenzione, perché noi in Italia siamo all'avanguardia e non si deve ritornare, durante il processo, che, se non c'è stato questo, significa che non è violenza sessuale, perché noi torniamo indietro. Noi, quando facemmo la legge, cambiammo il reato: ovviamente non un delitto contro la morale, ma un delitto contro la persona. Allora la persona, soprattutto durante il processo, deve essere tutelata tutelata nella sua dignità, sennò cominciamo a dire, come nella famosa sentenza: «Se hai i*jeans* stretti, vuol dire che sei stata consenziente: te li sei dovuti togliere». Roba, signor Presidente, che mi condannarono. Pensi, la Cassazione... Non le dico neanche quello che feci. Vabbè. Quindi, colleghi, concludo dicendo: benissimo questo dibattito. È fondamentale questa Convenzione, che deve essere di esempio a tutti e a tutte, e anche ai partiti politici, perché quello che stiamo vedendo quello che stiamo vedendo in alcuni partiti, dove si mandano via le persone con atti di violenza, senza che nulla succeda, è grossa. Anche questo dovrebbe essere inserito nella Convenzione. *(Applausi dai se la dovrebbe leggere. mi auguro veramente che ci sia la massima condivisione e che assieme alla ratifica, che - come diceva giustamente la collega Fattorini - poi dovrà essere accettata e ratificata da tutti gli altri Paesi, ci possa essere un adeguamento del nostro ordinamento, bello, cotto e mangiato, rapido, perché noi in Italia - ripeto - siamo all'avanguardia,

Sono presenti in tribuna gli allievi del Seminario di studi e ricerche parlamentari «Silvano Tosi» di Firenze, accompagnati dal professor Paolo Caretti.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ritengo di non esagerare nel dire che sono molto felice di intervenire per portare il mio modesto contributo all'approvazione della ratifica della Convenzione di Istanbul. Felice perché è uno dei primi provvedimenti di questa legislatura, e quindi destinato comunque a caratterizzarla; felice perché avviene in un Parlamento particolarmente rinnovato nelle presenze e in cui il segno più distintivo, e mi auguro anche più duraturo, di questo rinnovamento è costituito proprio dalla significativa presenza di neoelette; felice perché considero inderogabile che questa battaglia non resti solo confinata tra le giuste rivendicazioni delle donne, ma possa vedere accanto a loro tutti gli uomini possibili, a partire soprattutto da quelli che sono impegnati nelle istituzioni e che le rappresentano. Siamo rimasti indifferenti troppo a lungo. Dal Ratto delle sabine in poi abbiamo lasciato che la violenza contro le donne diventasse un vero e proprio massacro. Con il brutto termine femminicidio siamo oggi usi appellare quello strazio praticamente quotidiano che arma la mano degli uomini contro le proprie compagne. Le istituzioni non hanno ancora risposto adeguatamente, ecco perché probabilmente il massacro non si ferma. Le cronache ci parlano ogni volta di fenomeni non occasionali e mai estemporanei, ma episodi strutturati, talvolta premeditati con cura ed eseguiti con inimmaginabile freddezza. Episodi su cui è difficile intervenire perché anche preventivamente si alza spesso, proprio da parte delle ignare vittime, una cortina protettiva fatta di omertà e di paura, talvolta perfino di protezione nei confronti del proprio carnefice. Ora, si dice, è il momento della tolleranza zero. Ma perché questa affermazione non sia soltanto vuota retorica, occorre che a tolleranza zero corrisponda a mille il valore della prevenzione, altrimenti il rischio è solo quello di un vacuo proposito o di un editto di carta. La matrice culturale in cui si inquadra la quasi totalità degli episodi è quasi sempre la stessa, quella di un improprio senso del possesso, ancestrale o tribale che sia, per la sorella, la moglie, l'amata, l'amante, la donna, insomma, quale compagna altra da noi, a cui non si concede la pretesa, o la richiesta, sussurrata, gridata o implorata, il tentativo di un'autonoma libertà di parola, di pensiero, di sentimento o di amore, prima ancora che per l'altro, diverso da noi, per se stesse. È quindi un fondamentale aspetto di cultura e di rispetto, in una parola di educazione, a cui sistematicamente l'uomo manca. È il luogo delle mura domestiche, il luogo di protezione per eccellenza ad essere violato e profanato. Dietro gli scuri delle nostre case spesso si cela una sofferenza silenziosa, vite fatte di soprusi e di dolore inflitti a donne che non sono state ai patti, che sono uscite dal solco delle regole assegnate. L'assassino o l'aguzzino è quasi sempre il marito, l'amante o l'amato, tradito o rifiutato, allontanato o scoperto. In ogni caso, è sempre il gesto e l'azione cieca che sopraffà una relazione non più recuperabile con le parole e a cui la forza della violenza tende inesorabilmente per ristabilire sottomissione e dominio e, quando ciò non è più possibile, la soppressione appunto, nei modi e nelle forme più barbare. Ciò che più oltraggia è perfino la rimozione postuma del delitto: molti di questi infatti sono spesso taciuti o relegati a generici avvenimenti di cronaca. Non è più possibile accettare che tutto ciò continui a consumarsi sotto occhi indifferenti e orecchie distanti. Da domani, con la ratifica di questa Convenzione, dovrà essere chiaro che quando un uomo prende a botte una donna non costituisce un fatto privato o domestico perché consumato tra le quattro mura familiari. Da domani quelle botte e quegli urli chiamano in causa la nostra coscienza e interrogano il nostro grado civiltà. La Convenzione di Istanbul non è che un primo passo, una condizione necessaria, ma assolutamente non sufficiente. A partire da domani sarà indispensabile favorire davvero politiche di formazione per tutti coloro che sono coinvolti nell'accoglienza, nel recupero, nella difesa e nella tutela delle donne che subiscono violenza, una *task force* - è stato detto - che metta in rete le questure, i pronto soccorsi, gli studi legali, i tribunali, i centri antiviolenza. È necessario favorire la formazione di sezioni specializzate per l'organizzazione delle procure, in maniera tale da trattare in via prioritaria le situazioni di violenza. Occorre soprattutto la maturazione di una nuova coscienza con obiettivi culturali che si devono porre nelle scuole di ogni ordine e grado, dalla materna all'università, attraverso la stampa, in televisione e sulla rete. È stato importante e significativo, per il nostro Paese e per questo Parlamento, ratificare rapidamente questa Convenzione, ma se non vogliamo che tutto si riduca soltanto (anche se non è poco) a un bel gesto occorre dare continuità d'azione. Per questo chiedo ai Presidenti di Camera e Senato l'avvio immediato di una Commissione o di un Comitato (senza oneri per le Camere) che metta in rete le Commissioni giustizia, affari sociali, sanità, cultura, affinché in tempi certi stabilisca una lista di priorità, renda operative le leggi e ne predisponga controlli periodici sul suo effettivo stato di attuazione. Signor Presidente, signora rappresentante del Governo, colleghi senatrici e senatori, come senatrice, come persona impegnata nelle istituzioni, ed in primo luogo come donna, ho sempre avuto al centro del mio impegno politico, istituzionale e nella società civile il contrasto alla violenza contro le donne. Il femminicidio, gli omicidi della donna in quanto donna, ovvero gli omicidi basati sul genere, ovvero la maggior parte degli omicidi di donne e bambine sono un atto barbarico con cui tutti i giorni ci troviamo a confronto, nei volti e nelle storie di donne che avremmo potuto vedere accanto a noi nella vita di tutti i giorni e che invece troviamo purtroppo come terribili fatti di cronaca sui giornali. Si tratta di fatti violenti, di una violenza agghiacciante e terribile, immersi in una quotidianità di sopraffazione, disprezzo e mancanza di rispetto dei diritti umani; fatti ripetuti, a volte denunciati inutilmente, altre volte accettati come un male ineludibile, come un destino, ricordo - hanno portato alla morte nel nostro Paese 124 donne nel 2012: una strage e un continuo stillicidio, di cui purtroppo abbiamo consapevolezza solo quando una donna muore. Una violenza diffusa e continua infatti pervade la nostra società e viene considerata ordinaria. Questo è inaccettabile, e lo dobbiamo affermare con forza. Non dobbiamo dimenticare il dato riportato dalla «Casa delle donne», secondo cui il 40 per cento delle donne uccise in Italia lo scorso anno aveva già subìto violenze precedenti al femminicidio. Può essere un dato non corretto, ma certamente sono tante le donne uccise dopo aver subìto per anni violenza ed averlo denunciato. Questo, però, non è un destino; non sono un destino la violenza e la sopraffazione; non sono un destino i pregiudizi. colleghi, oggi in quest'Aula, con la ratifica della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, facciamo solo un primo passo per uscire da questa triste realtà, ma un passo importante. La Convenzione infatti riconosce la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione; stabilisce un chiaro legame tra 1'obiettivo della parità tra sessi e quello dell'eliminazione della violenza sulle donne. È un primo atto con cui ci si impegna tutti a risolvere un problema endemico della nostra società, anche promuovendo il cambiamento di comportamenti, incoraggiando gli uomini e i ragazzi a prevenire la violenza, vigilando perché la cultura, i costumi o la religione non siano utilizzati come pretesto per giustificarla, ma soprattutto promuovendo programmi e attività destinati ad aumentare l'autonomia e 1'emancipazione delle donne. È un atto con cui si pone al centro la vittima creando una forma di valutazione e gestione dei rischi e anche una più efficace azione punitiva. di evitare che si possano ripetere fatti come quelli descritti da Gian Antonio Stella sul «Corriere della Sera» di qualche mese fa. Ricordo, ad esempio, Emiliano Santangelo, che appena esce dal carcere, uccide la ragazza che lo aveva fatto condannare per violenza sessuale; Paolo Chieco, che, condannato a 12 anni, poi ridotti a 8 anni, per tentato omicidio della convivente Anna Rosa, ottiene i domiciliari a 300 metri dalla casa di lei e finisce di ucciderla; Luigi Faccetti che, condannato a 8 anni per tentato omicidio della fidanzata, dopo appena dieci mesi ottiene i domiciliari e la uccide con 66 coltellate. Queste norme di prevenzione, di protezione e di punizione (tre "p") sono importanti, e io sollecito qui il Parlamento, noi tutti perché, anche nelle more dell'entrata in vigore della Convenzione, si attuino queste misure. Sollecito anche il Governo perché si impegni a raggiungere in Europa il numero di ratifiche necessarie per l'entrata in vigore della Convenzione. La Convenzione è solo un punto di partenza, ma importante, perché la violenza viene finalmente riconosciuta come violazione dei diritti umani perché cita la prevenzione, la formazione e l'educazione come elementi per combattere questa violenza e per combattere la discriminazione di genere.

«I pregiudizi sono profondamente radicati nel costume: sfidano il tempo, le rettifiche, le smentite perché presentano un'utilità sociale. L'insicurezza umana ha bisogno di certezze, ed essi ne forniscono. (...) vengono trasmessi come verità indiscutibili fin dall'infanzia e non vengono mai rinnegati successivamente. L'individuo li interiorizza suo malgrado, e ne è vittima sia colui che li formula e li mantiene in vita contro l'altro, sia colui che ne viene colpito e bollato». Se riuscissimo, tramite l'educazione, mettere in luce questi pregiudizi e a rieducare le nuove generazioni a un rispetto delle persone, indipendentemente dal loro sesso, avremmo reso questo Paese migliore, migliore, non solo per le donne o le bambine, ma anche per gli uomini e per la società in cui viviamo.

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul 1'11 maggio 2011, è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La Convenzione riconosce un principio che dovrebbe essere ovvio: la violenza sulle donne è una violazione dei diritti umani. Interviene specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, come bambini e anziani, a cui si applicano le medesime norme di tutela. La rapida calendarizzazione del disegno di legge di ratifica denota un profondo impegno politico, che si intende perseguire anche in questa legislatura. Nonostante la gravità e la frequenza dei fatti di cronaca che riguardano la violenza sulla donne è bene evidenziare che, nel nostro Paese, le azioni di contrasto non partono da zero, ma che oggi occorre proseguire il percorso avviato nella XVI legislatura con l'introduzione del reato di *stalking* e delle aggravanti al reato di omicidio (alle donne è stato dato il patrocinio gratuito, tolto invece ai con il varo del piano nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking*, con il protocollo d'intesa siglato dall'allora ministro Carfagna con l'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria 26 gennaio 2011 per la tutela della dignità della donna e il non incitamento alla violenza nei messaggi pubblicitari e, non ultimo, con la presentazione del disegno di legge, a prima firma della senatrice Mussolini, recante l'introduzione di circostanze aggravanti nel femminicidio. Particolarmente rilevante è l'ampio spazio che la Convenzione dedica alla prevenzione, che richiede, innanzitutto, un profondo cambiamento culturale, perché le radici di questa violenza hanno una matrice culturale. Per tale ragione, accanto ai necessari interventi legislativi, è necessario promuovere campagne di sensibilizzazione, favorire nuovi programmi educativi e formare adeguate figure professionali, coinvolgendo tutti gli attori della società, a partire già dall'ambito scolastico. In ultima analisi, è necessario rafforzare il sostegno alle vittime e dei minori che siano stati testimoni di atti di violenza, con una rete organica a livello territoriale che sia omogenea su tutto il territorio e in grado di fornire l'adeguato supporto socioassistenziale, sia multidisciplinare che multiprofessionale,

è stato detto in un intervento poco fa. Ebbene, la violenza sulle donne ha un caro prezzo in termini di costi a carico della collettività, che in Italia non sono mai stati calcolati ufficialmente, come invece è stato fatto in diversi Paesi. Un calcolo sommario si deve al Consiglio d'Europa, che parla di 2,4 miliardi l'anno solo in Italia per far fronte al fenomeno e di 33 miliardi se si calcola la spesa annua sostenuta in tutto Il contrasto alla violenza richiede uno sforzo corale. Oltre all'intervento istituzionale con l'introduzione di misure legislative e un supporto adeguato, anche in termini di risorse, vorrei in questa sede lanciare un appello alla stampa e uno alla magistratura. Alla prima, per il modo in cui vengono veicolate le notizie. Quando leggo titoli come «Lei lo lascia e lui la uccide», sembra quasi che la donna abbia provocato il proprio carnefice, insomma, «che se la sia andata a cercare». È un messaggio pericolosamente distorto, che può contribuire a lasciare sommersi molti casi di violenza che si consumano tra le mura domestiche o tra gli affetti più intimi. Donne vittime o autrici di crimini. Quali termini utilizzano i *media* per descriverli? Può il linguaggio utilizzato influenzare il giudizio del pubblico? Credo di sì. Mi appello, inoltre, alla magistratura per chiedere tempi certi per perseguire questi gravi reati. Secondo i dati del Ministero della giustizia, nel 2010 la durata media delle indagini preliminari relative al dato di violenza sessuale, si sono concluse con un rinvio a giudizio, è stata di 373 giorni, circa 400 giorni, a cui si aggiungono più di 580 giorni per arrivare ad una sentenza di primo grado; quando va bene, più di tre anni. una mia riflessione; da mesi siamo minuziosamente informati su un processo a Milano, dove non c'è una vittima e non c'è una denuncia, ma il tempo intercorso tra le indagini preliminari e la sentenza di primo grado, attesa per il 24 giugno, è di dal Gruppo PdL)*. Una sentenza che sembra già scritta dall'inizio del processo, per come è stato condotto e, forse, anche per questo motivo, solo quattro italiani su dieci hanno dichiarato di avere fiducia nella giustizia. Mi viene in mente, al contrario di tutto ciò, che in un Comune del viterbese, Montalto di Castro, una ragazza, a sette anni dalla violenza di gruppo che ha subito da otto suoi coetanei, alla luce dei continui rinvii processuali, ha ritirato la denuncia e ha dichiarato: «se avessi saputo che finiva così, non li avrei mai denunciati», e di essere stanca e di non avere più la forza di combattere per la continua messa in prova degli aguzzini, ormai dall'epoca dei fatti ampiamente maggiorenni, senza poterli mai vedere, in sette anni, seduti sul banco degli imputati. Un'altra ferita inferta da una giustizia a rallentatore, che scoraggia le donne a denunciare, mentre in altri casi, ad esempio *ad personam*, ci sono delle accelerazioni sospette. Una spirale di dolore, che suscita la nostra indignazione, soprattutto al cospetto di notizie come quella relativa al delitto di Rubiera, in cui l'assassino, reo confesso dell'omicidio della compagna, è uscito dal carcere esattamente un anno dopo il delitto per decorrenza dei termini di custodia in pratica perché i magistrati non hanno trovato il tempo per fissare la prima udienza del processo. Alla luce dell'attuale scenario, credo che sia unanime la consapevolezza che la ratifica della Convenzione di Istanbul è solo il punto di partenza di un impegno ben più ampio che dovrà essere declinato nei provvedimenti e nelle sedi più opportune per arginare, in modo strutturale e non solo emergenziale, la violenza sulle donne.

è stato ribadito da tutti gli oratori che la violenza contro le donne è una violazione dei loro diritti, ed in particolare una violazione dei diritti umani. Le condotte sanzionate dalla Convenzione di Istanbul sono in gran parte già previste dal nostro codice penale, ma gli strumenti della tutela penale non sono sufficienti: va affrontata la dimensione culturale nella quale prolifera il clima di violenza contro le donne. Sono stata contenta, contentissima, di sentir parlare di prevenzione culturale proprio dal mio collega del Partito Democratico, il senatore Filippi. Tuttavia, un uomo solo in questo dibattito è insufficiente: voglio sentire la voce dei senatori su questo

settimane fa: dopo il quarto esposto una donna è stata uccisa dall'uomo che per quattro volte lei aveva cercato di far perseguire dall'autorità giudiziaria. Lascio a questo dibattito la conclusione, ma qualcuno dovrà pur far luce su questa inadempienza delle pubbliche autorità. Ora faccio un passo avanti e torno al testo della Convenzione di Istanbul, che identifica nel Ministero dell'interno il soggetto deputato a vigilare sull'attuazione della Convenzione. Sono previste campagne informative e l'istituzione di osservatori. Bene ha fatto la ministra Idem a proporre una *task force*, credo che però questo non sia sufficiente. Non è sufficiente, se non arriviamo a radicare nei territori, nei Comuni, nei luoghi dove si fa anche formazione una vera e propria cultura, partendo da esempi concreti. Penso alle buone pratiche: la collega Idem può trovarne

a una delibera, obbliga il sindaco a costituirsi parte civile al fianco delle donne vittime di violenza. Il Comune di Roma, inoltre, ha vietato la pubblicità lesiva della dignità della donna nei suoi spazi comunali. facciamo sì che le buone pratiche che le associazioni e tante consigliere comunali hanno imposto nei loro Comuni siano utilizzate dal Ministero.

Signor Presidente, non ho chiesto di intervenire perché sono un uomo e non una donna, ma per esprimere pochissime considerazioni. Mi è tornato in mente un dibattito al quale partecipai durante il conflitto nella ex Jugoslavia, in cui lo stupro fu utilizzato ai fini

Due brevi considerazioni. Ringrazio veramente la collega Fattorini per l'ottima relazione. Credo che la dobbiamo rileggere tutti, perché non è stata ascoltata come

tutti i giorni nella nostra attività di legislatori, ma anche nella società, di fronte a tutte quelle violenze che noi a volte vediamo senza intervenire. La legge non può risolvere tutto. La collega Fattorini ha parlato di sovraesposizione mediatica del tema. Vorrei parlare di un'altra sovraesposizione, anche se non so se un giorno si potrà legiferare su questo punto: com'è possibile continuare ad accettare che alcune trasmissioni televisive incentrate su atti di violenza gravi,

che, sfogliando le pagine, mostrava la giovane che è stata uccisa e bruciata viva da un coetaneo. Questa non è violenza? Per vendere qualche copia in più? Per qualche punto di *share* in più? Credo che la legge non basti, ma occorra la consapevolezza dei nostri doveri: noi come legislatori, ma anche tutti gli attori della società. Concludo dicendo che questo dibattito, caro

sulla situazione politica dei partiti attualmente in gioco in questa legislatura. Non credo che sia utile e all'altezza del dibattito che necessita questo tema.

Colleghi senatori, senatrici, signor Presidente, dal dopoguerra l'Italia ha vissuto una sorta di rinascimento, che ha permesso al suo popolo un'evoluzione vertiginosa sotto tutti i profili. Nella nostra società la lotta per la libertà, l'emancipazione e la parità sostanziale della donna risale agli anni Settanta, durante i quali vennero ottenuti grandi risultati per quanto riguarda l'autonomia della donna e la libertà di decisione sulla vita, sul lavoro e sulla maternità. Nel nostro Paese, in particolare, le tappe fondamentali sono state quelle del diritto al voto, nel 1946; della tutela delle lavoratrici madri, con la legge n. 1204 del 1971; la legge sul divorzio del 1970; le leggi sulla parità di trattamento tra uomini e donne e sull'interruzione volontaria della gravidanza, del 1977 e del 1978. Queste leggi, per cui ho lottato in prima persona durante quegli anni, mi hanno permesso di crescere in modo dignitoso i miei due figli e allo stesso tempo di condurre un'esistenza decorosa e libera. Negli ultimi anni, invece, sembra che la spinta riformatrice che ha alimentato l'emancipazione della donna si sia esaurita. Le donne, che erano riuscite nello scorso secolo, dopo molte battaglie e sacrifici, ad aver riconosciute le proprie capacità culturali, lavorative e sociali e a liberarsi da comportamenti discriminatori nei loro confronti, sono state colpite da una *escalation* di atrocità inconcepibile. Tutti i giorni le cronache ci informano di omicidi efferati, compiuti da mariti, conviventi o estranei, che a causa della perdita dell'oggetto del loro desiderio, o per follia pura, si accaniscono sui corpi di povere donne sventurate che non hanno la possibilità di difendersi. Stupri, acido, coltelli: la violenza si manifesta in ogni modo, e non solo da parte di soggetti provenienti da altri Paesi che appartengono ad una cultura diversa dalla nostra, come molto spesso i *media* vorrebbero farci intendere, ma anche da parte degli italiani stessi che sono cresciuti in condizioni ambientali più favorevoli. Sicuramente responsabile è l'abbassamento del livello culturale, dovuto ai pochi investimenti nella cultura da parte del Governo in questi anni e alla cattiva e alla cattiva informazione televisiva con un basso profilo culturale, che non fa crescere il livello di educazione a rapporti sociali equilibrati. Complice del mancato completamento dell'emancipazione femminile nel nostro Paese è stata anche la politica. Questo Parlamento, negli ultimi anni, non è mai stato esemplare nell'incentivare la dignità della donna. Anzi, alcuni comportamenti del nostro ex *Premier*, che non vedo mai hanno evidenziato che il trattamento riservato alle donne è stato sempre, sistematicamente, di svilimento e di degrado. E non sto parlando solo di infelici battute sessiste, che pure hanno costantemente colorito interventi e uscite pubbliche, ma del sistema vergognoso e dibattuto in ambito giudiziario che ci ha abituato a termini come «assaggio di ragazze» e «consumatore finale» Chi si è prestato a questo sistema per anni senza proferire verbo, utilizzando quest'Aula solo per fare *gossip*, invece che per battersi per il diritto delle donne, è considerabile in maniera ancora peggiore. È del tutto evidente che sottoscrivere una Convenzione che promuove la lotta contro la violenza nei confronti delle donne non basta a risolvere i problemi di mentalità del Paese, ma fondamentale deve essere l'esempio che proviene dalle istituzioni. Il pericolo che la Convenzione di Istanbul diventi un guscio vuoto, se non accompagnata da un radicale cambiamento culturale, non è remoto: basti pensare che tra i primi Paesi che l'hanno ratificata vi è anche la Turchia che, come abbiamo avuto modo di osservare negli ultimi tempi, sta praticando politiche retrograde che tendono a riportare la condizione della donna indietro nel tempo, con la minaccia di introdurre leggi per vietare l'aborto e i metodi contraccettivi. Si ha la sensazione che in quel Paese la ratifica della Convenzione sia stata usata in modo del tutto ipocrita per mettere a tacere i rimproveri dell'Europa, ma senza la vera volontà di attuarla in maniera concreta. Tale pericolo deve essere scongiurato nel nostro Paese ed alla ratifica della Convenzione di Istanbul deve seguire un percorso normativo di attuazione e di educazione alla cultura del rispetto della donna. Il mio è un grido di dolore per tutte quelle giovani, e non più giovani, donne a cui è stata negata la possibilità di vivere la loro vita. E la cosa che più mi indigna è che, per molti di questi assassini e aguzzini, il sistema giudiziario infligge condanne lievi, lasciando così che molti si ritengano autorizzati a perpetrare ulteriori efferatezze. *(Applausi dal

la Commissione bilancio, alla quale appartengo, è stata chiamata ad esprimere il parere rispetto al disegno di legge di ratifica della Convenzione, e si è così espressa: parere non ostativo, ma con la raccomandazione di dare copertura ai provvedimenti attuativi. È evidente che gli articoli 2 e 3 del disegno di legge non sono coerenti fra di loro: non è credibile la volontà di dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione prevedendo contemporaneamente la clausola di neutralità finanziaria che prevede che «le misure amministrative necessarie all'attuazione e all'esecuzione della Convenzione sono assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». Questa clausola sarebbe estremamente positiva e all'avanguardia se fosse l'espressione dell'accoglimento della logica dei bilanci di genere, ovvero di un'attenzione trasversale alle tematiche di genere: questo vorrebbe dire che tutti i settori della pubblica amministrazione sono orientati e sensibili al riequilibrio. Ne prendo atto, pensando che da oggi carabinieri, forze dell'ordine, sanità, scuola sono magicamente orientati ad una riallocazione delle risorse per una prima risposta di applicazione della Convenzione. Esempio positivo di questo approccio trasversale è stato l'inserimento nel decreto svuota carceri di due punti della Convenzione: un osservatorio di analisi di criminologia sulla violenza di genere e, cosa ancora più importante, la possibilità di ottenere lo *status* di residenti, indipendentemente dal *partner*, per le donne emigranti soggette ad abusi e persecuzioni. Quindi, c'è stata un'attenzione del genere all'interno di un provvedimento generale. Ma questo è possibile per tutte le politiche previste dalla Convenzione di Istanbul? La Convenzione, nell'articolo 1, impegna lo Stato a predisporre un quadro globale di politiche e misure di protezione di tutte le vittime. Tra le molte politiche ne prendo ad esempio una sola, la realizzazione delle case rifugio prevista dall'articolo 23: le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare alle donne e ai loro bambini, e per aiutarle in modo attivo. In Italia ci sono 127 centri, di cui solo 61 sono delle vere e proprie case rifugio, per un totale in tutto il territorio del Paese di 500 posti letto. L'Unione europea raccomanda un centro antiviolenza ogni 10.000 abitanti, un centro di emergenza ogni 50.000 e 5.700 posti letto nelle case rifugio per uno Stato come l'Italia: un impegno economico ed organizzativo più che decuplicato rispetto all'attuale, soprattutto se si considera che attualmente la maggioranza delle case è gestita da associazioni di donne pressoché volontarie, con pochi aiuti da parte di qualche ente locale e qualche contributo privato.

In questo contesto va anche ricordata la bella campagna della Chiesa valdese, che dedica tutto il suo otto per mille alle donne maltrattate e perseguitate. Pensare però di rispettare questo obbligo senza risorse mi pare francamente impossibile. Mi sento di condividere quanto chiesto oggi da Mariella Gramaglia su «La Stampa» alle Ministre della*task force*: integrare questa legge "secca", come si suol dire in gergo parlamentare, ovvero senza finanziamento, con un progetto di fattibilità economica. Con una legge vera,

Signor Presidente, ringrazio la senatrice Fattorini e tutte le colleghe e i colleghi intervenuti

Convenzione di Istanbul consiglia a tutti gli Stati - non diventano atto normativo e non interviene il legislatore a trasformarli in norme,

dove più ampia ed equilibrata è la presenza delle donne. Tutte insieme dobbiamo dare forza alla Convenzione e alla Ministra per le pari opportunità, insieme alla *task

stanno lavorando per dotare il nostro Paese di un codice deontologico dei *media*, i quali spesso presentano i casi di femminicidio come frutto di delitti passionali. Desidero ricordare che il nostro è un Paese in ritardo, che agisce sempre con grave ritardo: il delitto d'onore è stato abrogato solo nel 1981. È per questo motivo che continuiamo ad utilizzare, anche nella rappresentazione pubblica, un linguaggio completamente sbagliato. Chiedo al Presidente del Senato, quindi, di calendarizzare al più presto, in Commissione giustizia, i tanti testi di legge presentati contro il femminicidio. Possiamo lavorare insieme e in Commissione avviare

calendarizzando i disegni di legge che abbiamo depositato, per dotare il nostro Paese di un testo all'avanguardia che si ispiri proprio alla Convenzione che stiamo ratificando.

Signor Presidente, colleghi senatori, prima di tutto permettetemi di ringraziare tutti quegli uomini - e ce ne sono molti, per fortuna - che ogni giorno dimostrano nei fatti il loro rispetto nei confronti delle donne. Sembra assurdo dover ringraziare per qualcosa che dovrebbe essere invece scontato, naturale e dovuto. Eppure, oggi sono ancora troppi gli uomini che pensano alle donne (mogli e figlie, soprattutto) come ad una proprietà, un bene di cui disporre a proprio piacimento e che, quindi, può essere sfruttato e maltrattato. E così ci ritroviamo, nel terzo millennio, ad avere la necessità di discutere mozioni e di affrontare ratifiche volte a prevenire e ad arginare la violenza nei confronti delle donne, e soprattutto la violenza domestica. Gli interventi da un punto di vista legislativo sono importanti e la parità di genere tra uomini e donne deve essere garantita e ribadita in tutte le sedi istituzionali.

ma mi permetto di dire che non è abbastanza. Questi interventi devono essere accompagnati, sostenuti e avvalorati da un concreto cambiamento a livello culturale, La violenza sulle donne - e più in generale la violenza domestica nei confronti dei bambini e degli anziani - deve essere considerata aberrante da tutti, è un colpo al cuore per l'identità profonda della famiglia e della società. Proprio per questo, con la mozione n. 56 chiediamo anche che vengano messe in atto iniziative volte a promuovere la conoscenza e l'applicazione effettiva della normativa vigente in tema di tutela dei diritti umani e di contrasto alla violenza sulle donne, in particolar modo attraverso la promozione di un programma di educazione che deve partire fin dalle scuole

che anche in quelle società cosiddette avanzate, che fanno un vanto del tema dei diritti civili e di parità di genere, molto spesso accadono episodi di violenza di genere.

Un'indagine del 2006 riporta che il 32 per cento delle donne tra i 16 e i 70 anni è stato fisicamente o psicologicamente abusato durante la propria vita (una su tre), ma solo il 18 per cento delle donne che hanno subito violenza lo considera un crimine. Si stima che tuttora il 90 per cento degli abusi, compresi gli stupri, non venga denunciato. La Convenzione di cui oggi discutiamo individua anche una serie di reati - tra cui la violenza psicologica, l'aborto forzato, le molestie sessuali, il matrimonio forzato - che gli Stati si impegnano a introdurre qualora non siano già presenti

Una donna che subisce queste violenze deve compiere uno sforzo enorme per riuscire a sporgere denuncia, e non lo farà se l'azione penale è quasi nulla. *rapportenz* dell'ONU Rashid Manjoo evidenzia che l'ulteriore danno alle donne è rappresentato dai ritardi della giustizia, che rendono inapplicabili le sentenze di condanna

poi è stata accusata di avere istigato la violenza con il proprio abbigliamento troppo provocante. La questione culturale è centrale e richiede una rivoluzione profonda per sradicare gli stereotipi di genere, che nel nostro Paese sono ancora così radicati. Si deve arrivare ad un cambiamento culturale profondo, ma è necessario partire da salvaguardie a livello ordinamentale. Sotto questo profilo, il nostro Paese è certamente tra quelli che maggiormente garantiscono quanto richiesto dalla Convenzione che oggi ratifichiamo. Le misure legislative ed amministrative adottate negli ultimi anni sono state dei passi importanti. Ricordiamo, ad esempio, le norme ricomprese nell'ambito dei delitti contro la libertà morale, volte a punire chiunque comprometta l'integrità psicologica di una persona con la coercizione e le minacce; la norma volta a punire la commissione di atti persecutori; le norme ricomprese nell'ambito dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale, volte a penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona. Eppure, nonostante tutte queste norme, negli ultimi mesi abbiamo letto con troppa frequenza sulle pagine di cronaca episodi di violenza grave e gravissima contro le donne. La parola "femminicidio" è entrata nell'uso comune e questo può forse dare l'impressione che il fenomeno sia improvvisamente esploso. I numeri, a dir poco allarmanti, confermano che gli eventi di questo genere sono numerosi, ma non sono certo un fenomeno odierno. Il fatto che se ne parli, che ci sia una condanna unanime della mentalità dispregiativa alla base della violenza, che si prenda coscienza dei fenomeni di femminicidio non basta se poi le donne continuano a subire ad intervalli costanti pressioni fisiche e psicologiche, ma è certamente importante per avviare un dibattito onesto sul tema e per trovare coralmente il modo di porre fine a questi crimini. La Convenzione torna in più punti sull'inaccettabilità di motivazioni fondate sul «la cultura, gli usi e i costumi, religione, sulle tradizioni o sul cosiddetto onore a giustificazione delle violenze, chiedendo agli Stati di introdurre, anche qui, misure legislative atte a contrastare i fenomeni di violenza. Pensiamo, ad esempio, al matrimonio imposto dalla cultura dei musulmani presenti in Italia, come il caso di quella ragazza uccisa dal padre solo perché si era fidanzata con un ragazzo italiano. O alla tradizione della mutilazione dei genitali femminili, diffusa anche qui in Italia, cosa a nostro parere gravissima. parere gravissima. O al velo, che spesso le donne di diversa etnia sono obbligate ad indossare contro la loro volontà, spesso imposto con la minaccia, che lede la dignità delle donne e rappresenta una forma dì violenza. Nel nostro Paese negli ultimi dieci anni il numero complessivo degli omicidi è diminuito, ma il numero degli omicidi perpetrati nei confronti delle donne è aumentato in maniera preoccupante (i dati relativi al 2012 in Italia registrano più di 120 vittime). E spesso queste violenze, purtroppo, nascono nel cuore delle relazioni e della vita familiare. Sono tante, troppe! È importante parlarne, ma ancora più importante è continuare a sconvolgersi ogni volta: sarebbe catastrofico cominciare ad abituarsi all'idea che succeda. Non può diventare uno di quei fenomeni eccessivamente evocati e condannati, che rischiano paradossalmente di rendere assuefatti. Questo trattato ha un alto valore simbolico per il Parlamento e per il Paese: il Parlamento si è adoperato per recepire coralmente, e con la massima tempestività questo documento del Consiglio d'Europa, che non stravolge l'architettura giuridica del nostro ordinamento, ma certamente vorrebbe avviare una rivoluzione culturale, perché pone il problema in primo piano tra le emergenze a cui rispondere. Assemblea ha voluto affiancare anche altri impegni: quelli previsti dalle mozioni oggi in esame. Si vuole quindi affermare chiaramente che questa che questa odiosa forma di violenza intendiamo riconoscerla e non fare finta di niente; vogliamo condannarla, senza eccezioni, così come vuole la stragrande maggioranza dei nostri concittadini. Mi permetto di aggiungere anche che la nostra mozione cerca di perseguire il programma diretto a contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, promuovendo il sostegno, anche attraverso appositi finanziamenti, della rete dei centri antiviolenza presenti sul nostro territorio nazionale. Oggi discutiamo di queste mozioni e di questa Convenzione perché vogliamo trovare degli strumenti che affrontino il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica in modo completo, riservando il giusto spazio sia a strumenti legislativi che processuali, compresa l'assistenza processuale e i servizi di supporto specializzati, nonché alla prevenzione, alla sensibilizzazione, all'educazione e all'informazione. L'impegno è che le disposizioni di tutela dalla violenza contro le donne vengano applicate sia in tempo di pace che in tempo di guerra, ben sapendo tutti che durante i conflitti le regole saltano e i comportamenti più aberranti dilagano. La Lega Nord voterà convintamente a favore della ratifica della Convenzione e degli impegni chiesti nelle mozioni per contrastare la violenza sulle donne. c'è ancora tanto da fare perché la parità di genere, riconosciuta dalla Costituzione, venga vissuta veramente anche nel quotidiano di tutti noi. Salutiamo una delegazione della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Innsbruck, in Austria.

Signora Presidente, rappresentante del Governo, care colleghe e cari colleghi, come è stato sottolineato da tutti gli interventi che mi hanno preceduto - e in particolare mi sento di ringraziare la relatrice, senatrice Fattorini -, la Convenzione di Istanbul è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante vincolante che stabilisce come violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione la violenza sulle donne. Sappiamo, attraverso i dati forniti da organizzazioni internazionali, europee e nazionali, che la violenza sulle donne è agita prevalentemente in ambito familiare, particolarmente dai *partner* conviventi o ex conviventi, ed è la prima causa di morte per le donne dai 16 ai 50 anni, in Europa e nel mondo, e nel nostro Paese lo è più che in altri. Sappiamo come la violenza sulle donne attraversi tutti gli strati sociali e sappiamo che non è espressione quasi mai dello scarso livello culturale, ma è certamente la drammatica conseguenza del permanere nella nostra società di stereotipi e pregiudizi sui ruoli delle donne e degli uomini. La drammatica crescita di atti di violenza contro le donne ha reso necessaria la nascita di una nuova parola. È stato necessario trovare il termine che ne significasse immediatamente l'efferatezza e l'odiosa, drammatica specificità; è stata questa urgenza che ha portato le donne a coniare il termine "femminicidio". Le colleghe e i colleghi che mi hanno preceduto hanno detto moltissimo delle questioni fondamentali che la Convenzione traccia negli impegni dei Paesi che la ratificano, quindi vorrei soffermarmi su un aspetto specifico che attiene all'ambito vasto della prevenzione e a quello dell'accoglienza delle vittime che riescono a fuggire dalla violenza. La Convenzione ci chiama a mettere in atto la lotta contro la violenza di genere attraverso politiche di prevenzione, di protezione, di repressione, e ci chiede di monitorare il livello dell'integrazione delle singole politiche. penso vada potenziata la formazione specializzata ed integrata di tutti gli operatori sociali, sanitari e giudiziari che incontrano le donne in concomitanza con le violenze subite e che consente di intraprendere con le stesse un percorso di recupero psicologico e soprattutto di riacquisizione della piena propria identità. Per questo credo che sia importante promuovere e sostenere, anche economicamente, processi di formazione interprofessionali e interistituzionali che favoriscano il riconoscimento di azioni e linguaggi comuni. Sappiamo purtroppo che tante vittime, ma anche tanti carnefici, sono giovani, spesso adolescenti. Pensiamo che la prevenzione passi soprattutto attraverso il cambiamento di modelli culturali stereotipati e che la scuola uno degli ambiti fondamentali su cui lavorare per promuovere una diversa cultura di genere. Alla scuola però non possiamo affidare solo responsabilità, ma dobbiamo fornire anche supporti. Per questo chiedo che si ragioni sulla possibilità di istituire presso le scuole sportelli di accompagnamento psicopedagogico aperti all'accoglienza dei ragazzi, degli insegnanti e delle famiglie. Vi sono in questo senso preziose esperienze in tante scuole del nostro Paese, spesso promosse dagli enti locali, che sarebbe utile - io penso necessario - diffondere

Signora Presidente, colleghi, c'è un terreno fecondo su cui la democrazia si costruisce e si consolida ed è il terreno dei diritti e delle libertà, sociali e soggettive. È dovere della politica far sì che questo terreno sia ampio, aperto, inclusivo, evitare che il perimetro diventi muro invalicabile di diritti negati, riducendo la democrazia a parola vuota, senza significato. Ci sono oggi, nel secolo della democrazia, barriere che troppo spesso costringono le giovani generazioni e le donne in una condizione di anomia e minorità: fratture sociali, mancanza di lavoro, mancanza di diritti e tutele, di strumenti per emergere e per far valere il proprio talento nonostante e a prescindere dal luogo in cui si è nati e dalle condizioni in cui si è cresciuti. Nell'ultimo trentennio l'ideologia della diseguaglianza ha potuto configurarsi come modello sociale egemone, precipitando le società occidentali in una crisi che a sua volta genera e amplifica disparità e discriminazioni. Nel regresso della nostra società e della nostra democrazia c'è un interstizio di enorme gravità materiale e simbolica, la sequela della violenza di genere, una lunga e insopportabile cicatrice che sfigura il volto e l'anima della nostra Repubblica; violenza psicologica e fisica, fino al femminicidio, tanto più profonda perché perpetrata per lo più in ambito familiare o affettivo. Michelle Bachelet, in una bellissima testimonianza, ha ricordato un detto di quando era ragazza in Cile: «chi ti ama ti picchia». È un detto purtroppo familiare anche a noi, che rievoca il retaggio ancestrale di vincoli feudali mai del tutto sconfitti né sopiti, che anzi riemergono in questi anni di crisi, di ripiegamento, di insicurezze e di paure che travolgono certezze, identità e ruoli di ognuno. Nella mano che si scaglia, nel coltello che recide, nell'acido che corrode e nella violenza che insulta la donna c'è il tentativo di zittire una voce, di sopprimere una soggettività. Molto spesso la libertà è l'autodeterminazione più intima, estrema, talvolta dolorosa, che ognuno di noi ha: quella di dichiarare finita una storia d'amore, di sciogliere un vincolo familiare. Sta qui, nella sua portata antropologica, la forza emancipatrice della rivoluzione femminile, del pensiero della differenza, che è quintessenza della democrazia, che solo quando promuove cittadinanza ed inclusione può vincere populismo ed antipolitica. Ogni volta che una donna viene colpita, in un patetico tentativo di restaurazione simbolica di una gerarchia virile, è la democrazia ad essere colpita, oggi noi stabiliamo che questo sia il più infamante tra i crimini poiché vìola i diritti umani e nega la possibilità di un nuovo umanesimo, alla base di una nuova convivenza, una nuova educazione civile, il valore del riconoscimento reciproco, dell'autonomia rispetto al conformismo degli stereotipi in cui la mercificazione finanche dell'immaginario ha nuovamente ingabbiato uomini e donne. Violenza e democrazia sono una radicale antinomia. Istanbul, dove è stata siglata la Convenzione, da giorni è teatro di grandi manifestazioni. Gli alberi di Gezi Park sono divenuti per tantissimi, in Turchia, in Europa e nel mondo, emblema di libertà, da non sradicare. C'è un'immagine simbolo della protesta: una giovane donna, vestita di rosso, colpita con violenza dal getto di un idrante. Ecco, a quella giovane donna vanno le parole che Nazım Hikmet dalla prigionia dedicò alla compagna: «Verrà un giorno che gli uomini si guarderanno l'un l'altro fraternamente con i tuoi occhi». Avere gli occhi di chi subisce violenza, di chi è costretto ai margini, è nostro dovere in quest'Aula, oggi e sempre.

la ratifica della Convenzione di Istanbul rappresenta un deciso passo in avanti che il nostro Paese compie nella lotta alla violenza di genere e nel rafforzamento della tutela dei più deboli, in particolare delle donne, e che va ad affiancare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale, anche conosciuta come Convenzione di Lanzarote, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 12 luglio 2007. Tuttavia mi preme qui ricordare che a questo passo in avanti dovranno seguirne necessariamente altri, forse i più ardui, affinché quanto stabilito ad Istanbul non rimanga lettera morta. È infatti di vitale importanza che vi sia uno sforzo congiunto per trasformare le parole della Convenzione in azioni concrete, che costituiscano un'effettiva protezione per donne e bambini vittime di violenza ed abusi. La drammaticità e la tragicità degli eventi degli ultimi anni ce lo impongono. A tal proposito, credo sia assolutamente necessario, secondo diverse e concorrenti linee direttive, direttive, introdurre le opportune modifiche al nostro codice penale, in particolare per quanto concerne le parti relative ai maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (articolo 572 del codice penale), alla violenza sessuale (articolo 609-*bis* del codice penale) o alle circostanze aggravanti in caso di violenza sessuale (articolo 609-*ter* del codice penale), colmando così i vuoti legislativi, dove ve ne fossero, e perfezionando ed arricchendo la legislazione vigente.

in tal senso, che spero venga appoggiato). Se la norma, la mera norma, non è seguita da mezzi e strumenti concreti per poterla applicare, da sola non è uno strumento sufficiente. Dobbiamo impegnarci affinché chi è vittima di abusi venga inserito in un contesto di reale tutela. Occorre pertanto rilanciare strumenti come il Fondo per la realizzazione di un piano contro la violenza alle donne, creato presso la Presidenza del Consiglio con la legge finanziaria del 2008, che vede nella realizzazione che vede nella realizzazione di una rete nazionale antiviolenza il suo punto cardine e il cui scopo precipuo è di incentivare l'azione di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere e di promuovere la costituzione o il rafforzamento di reti locali atte a contrastare gli episodi di violenza e di *stalking*. Riteniamo inoltre sia imprescindibile che le forze dell'ordine siano effettivamente messe in condizione di intervenire tempestivamente ed efficacemente in caso di abusi nei confronti delle donne e, in particolare, in caso di *stalking*, fornendo loro gli strumenti necessari e snellendo le procedure burocratiche che guidano i loro interventi. Riteniamo infine di fondamentale importanza avviare dei percorsi di recupero per chi questi reati li compie, in quanto la mera pena detentiva in sé non costituisce uno strumento sufficiente a combattere una piaga così grave come il femminicidio. Manifestiamo quindi il nostro impegno per far sì che la Convenzione di Istanbul non segua lo sfortunato destino di altre Convenzioni internazionali che l'hanno preceduta in breve tempo un efficace e duraturo strumento di tutela. Il percorso è ancora lungo. La lotta contro la violenza di genere è solo agli inizi e non si può pensare che quello legislativo sia l'unico mezzo da utilizzare. È necessaria infatti una vera rivoluzione culturale, partendo proprio da noi uomini. Crediamo però che un corretto recepimento all'interno del nostro ordinamento di quanto disposto dalla Convenzione sia un passaggio imprescindibile affinché si avvii un reale cambiamento e a questa intollerabile situazione venga finalmente posto un efficace freno.

la Convenzione di Istanbul che ci apprestiamo a ratificare e sulla quale sono già ampiamente, e con dovizia di particolari, intervenute autorevoli colleghe senatrici - fortunatamente, anche colleghi senatori - a partire dalla relatrice Fattorini, rappresenta il primo strumento internazionale in grado di vincolare giuridicamente gli Stati alla tutela dei diritti delle donne. L'obiettivo è quindi quello di dar vita finalmente ad un quadro normativo completo, capace di contrastare e prevenire qualunque tipo di violenza contro le donne e quindi di predisporre un quadro globale di politiche e di misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza, in modo tale da mettere le autorità competenti in grado di agire e di collaborare efficacemente anche a livello internazionale. La Convenzione obbliga dunque gli Stati aderenti ad adottare tutte le misure legislative necessarie per la tutela delle donne vittime di violenza. Voglio ricordare a tutti che il Parlamento europeo, la scorsa settimana, riunito in seduta plenaria a Strasburgo, ha approvato una risoluzione sulla lotta al crimine organizzato. Le tradizionali organizzazioni criminali negli anni hanno progressivamente esteso il loro raggio di azione a livello internazionale, ed è oggi prioritario individuare gli strumenti legislativi per mettere in atto una strategia di contrasto effettivo alla pratica di tali cartelli mafiosi. Faccio questo inciso perché, all'interno della discussione dell'argomento all'ordine del giorno e relativamente ai contenuti

seria su un fenomeno sociale complesso quale quello della prostituzione. Credo che il nostro Paese oggi debba dotarsi di una legge che regolamenti l'esercizio della prostituzione, andando oltre la cosiddetta legge Merlin del 1958, obsoleta ed inadatta rispetto ai contesti nella quale si consuma oggi la prostituzione, anche se quella legge era nata da una giusta reazione alla politica regolamentarista del tempo, che violava i principi di eguaglianza e le libertà individuali. Una regolamentazione in tal senso è necessaria perché non regolamentare o, peggio, criminalizzare o proibire produrrebbe solo una sostanziale indifferenziazione tra libere scelte di autodeterminazione e prostituzione coatta, sfruttata, gestita dalle organizzazioni criminali di tutto il mondo, che gestiscono la tratta delle donne, soprattutto minori, sfruttandole, soggiogandole e sottoponendole a violenze indicibili attraverso l'impiego della minaccia, della forza e di altre forme di coercizione. Il fatto che lo Stato preferisca la non regolamentazione non è sicuramente orientato a privilegiare le prostitute, ma piuttosto a tutelare la *privacy* dei clienti e alla protezione omertosa del giro di affari illegali che la prostituzione alimenta. Auspico, quindi, che a partire da oggi, dopo la ratifica della Convenzione quale strumento internazionale, il Parlamento si faccia carico di aprire una seria e proficua discussione sull'argomento.

il tema della dignità della persona e dei diritti delle donne intesi come diritti umani ha conseguenze pratiche non irrilevanti. Innanzitutto, diritto umano significa benessere inteso come unione di benessere fisico e psichico. Non è accettabile che si parli ancora oggi di violenza contro le donne solo ed esclusivamente quando avviene quando avviene un fatto di violenza fisica. Credo che la violenza morale nei confronti delle donne, la persecuzione, lo *stalking* e l'insistenza siano paragonabili a pieno titolo ad una violenza fisica. Dico questo perché il primo problema che è certamente di tipo culturale, ma dobbiamo sapere anche che la violenza alle donne non conosce classi sociali sociali e latitudini. Come sapete, la violenza sulle donne ogni anno fa più morti del cancro e degli incidenti stradali e non sopporta e non può sopportare forme di relativismo etico. È per questo che, non a caso, la Convenzione di Istanbul, il tema delle migranti, che sono oggi oggetto di violenza, in modo rilevante anche nel nostro Paese, anche perché - diciamo la verità - dal punto di vista della tutela sanitaria, queste migranti sono molto spesso sorelle che non hanno hanno un diritto ed un accesso di cittadinanza, e provengono da culture per le quali è difficile uscire da sole di giorno e andare, non dico a denunciare, ma addirittura a farsi visitare da un ginecologo. È un tema straordinariamente grande perché ha a che fare con il significato della famiglia, dell'amore, della coppia e anche con quella struttura familiare, che appunto non ha latitudini e non conosce la diversità delle etnie culturali,

l'amore e la responsabilità di se stessi nei confronti dell'altro: temi davvero giganteschi. Può darsi che le leggi non siano tutto, anzi certamente non lo sono, ma senza le leggi non avremmo mai avuto quella crescita culturale che ha portato nel nostro Paese ad un grande avanzamento di civiltà sul piano del rispetto e del riconoscimento della libertà delle donne, della libertà nel rispetto del proprio corpo e dell'intangibilità del corpo femminile, se non dietro una scelta consapevole di una donna, della libertà nelle relazioni umane, della libertà anche per cose banali che sono oggi negate, come il poter uscire tranquillamente di notte senza avere la paura di tornare a casa e di venire aggredite. Anche di questo tema dobbiamo parlare,

credo che sarà consegnato solo ed esclusivamente alla pratica penale e al carcere. Credo che - secondo il «diritto mite» - ci sia bisogno della certezza della pena, ma anche della riabilitazione.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di intervenire perché credo che questo sia un tema di tutti, non solo di una parte, e che non ci sia una parte del cielo che deve intervenire per dimostrare sensibilità nei confronti dell'altra.

di mentalità, di clima, di cultura, di messaggio che viene trasmesso dalle televisioni e non solo e che alimenta questo fenomeno

infatti, che le nuove generazioni assumano una diversa sensibilità su questo tema se non cambiamo il tipo di messaggio, se non le formiamo in modo libero, laico e consapevole ad una responsabilità,

tra femminicidio e crisi della famiglia e dei nuclei conviventi, perché tutto quello che avviene, in termini di violenza alle donne all'interno della famiglia o dei rapporti di convivenza, è un messaggio disastroso per i figli e per la società.

secondo comma, della Costituzione, concernente il tema dell'uguaglianza sostanziale, per rimuovere un ostacolo che, di fatto, si frappone al pieno sviluppo della personalità femminile, ma - vorrei dire - anche della società nel suo complesso. Una società civile, infatti,

adeguato significa essere incapaci di dare quel segnale di repressione di certi fenomeni, che è importantissimo per essere credibili sul piano delle affermazioni di principio e sul piano della legislazione, che deve garantire il superamento di questa barbarie. *(Applausi Signor Presidente, ci stiamo occupando del fenomeno che si è preso a chiamare "femminicidio" non perché nel nostro Paese - dove certamente vi è una situazione molto diversa da quella di molti altri Paesi, anche di quelli che hanno firmato la Convenzione di Istanbul e, a maggior ragione, di quelli che non l'hanno fatto (ed è

donne che vengono uccise proprio in quanto donne, in quanto vittime di un atteggiamento di sopraffazione da parte di alcuni.

gli uomini in generale, ma soprattutto quelli che commettono questi reati, hanno da imparare dal comportamento generale delle donne, anche confrontando Pertanto, è importante isolare, dal punto di vista concettuale, il fenomeno dell'uccisione di donne in quanto tali, perché, in in alcuni casi (naturalmente non in qualunque assassinio di donne), esso è indice di un atteggiamento di sopraffazione, che a volte implica violenze di altri tipi, che sono certamente più numerose Tuttavia, bisogna anche evitare di confondere il patologico con la situazione la situazione generale della nostra società. Francamente non credo che in Italia ci sia costantemente e dappertutto un clima che favorisce e che in qualche modo giustifica e incoraggia un

Abbiamo un numero di omicidi inferiore anche a quello di molti di quei Paesi che hanno, sul piano della parità dei diritti tra gli uomini e le donne, una situazione storica più consolidata della nostra. Bisogna anche evitare atteggiamenti propri di uno Stato troppo pedagogico. Trovo degli esempi proprio nel preambolo di questa Convenzione, il cui testo ritengo sia per intero non non solo da accettare, ma sottoscrivibile e fortemente sostenibile. Nel preambolo ci sono delle espressioni che sicuramente possono essere valide in altri Paesi, ma francamente avrei davvero difficoltà nel caso del lo stesso. Si legge, per esempio: «Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini». uomini». Non penso che nel nostro Paese le donne siano costrette a una situazione sociale subordinata agli uomini, ma di certo, se ci sono delle situazioni

di questi documenti e, in particolare, dal substrato culturale che li ispira, credo vada preso con prudenza. Un'altra parte del preambolo Un'altra parte del preambolo si riferisce a rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione, e rileva che tutto questo si manifesta

direi che anche questa espressione è difficile da sostenere per il nostro Paese. Credo che dobbiamo evitare di sposare per intero filosofie che sono, per certi versi e da un punto di vista strettamente culturale, un po' estremistiche. Detto questo, è

sembrano prendere come assioma il concetto che la violenza sulle donne è un portato dell'antica società - dove indubbiamente c'erano ruoli molto diversi e, tendenzialmente, una subordinazione della donna rispetto all'uomo - e l'unico antidoto a questa violenza è la totale uomo e donna non soltanto dal punto di vista della legge - e ci mancherebbe: ce l'abbiamo nella nostra Costituzione da 65 anni - ma anche

che presupponga un ruolo subordinato della donna rispetto all'uomo e di qualunque stereotipo di specificità della donna rispetto all'uomo. In altre parole, non si potrà neanche più dire che una donna fa meglio

PSI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, ho chiesto e concordato con il Presidente della nostra Assemblea di avanzare una questione che avrei voluto fosse pregiudiziale, ma che discutiamo in questa fase dei nostri lavori. Si tratta dell'espulsione della senatrice Adele Gambaro, rea di aver rilasciato un'intervista ad una televisione privata.

Non è un fatto privato; non appartiene alla vita interna di un partito, ancorché, se vi appartenesse, sarebbe comunque emendabile, anzi condannabile. *(Applausi La mia opinione, signor Presidente, è che venga lesa una libertà costituzionale fondamentale, la libertà di pensiero, nell'espulsione da un Gruppo parlamentare e non da un partito si segni una svolta significativa. I Gruppi parlamentari da una parte della giurisprudenza italiana sono considerati alla stregua dei partiti. Conosco bene la polemica che nel tempo si è innescata e conosco, per averla studiata nel corso della notte e questa mattina, la polemica che nel tempo si è costruita: Gruppi ritenuti da una certa giurisprudenza simili a partiti. Io appartengo invece al ramo di chi ritiene che i Gruppi parlamentari non abbiano la natura dei partiti. I Gruppi parlamentari sono espressione di una struttura parlamentare. Sono infatti Gruppi parlamentari. Nella loro costituzione rispondono a regole. Se quelle regole non vengono rispettate, lei correttamente, signor Presidente, applicando la normativa, non consente la costituzione di un Gruppo, come la sua stessa collega Presidente della Camera non lo consente alla Camera dei deputati. Qui siamo addirittura di fronte ad un caso ancora più particolare, perché siamo in presenza di una sorta di censura,

signor Presidente, e ai nostri colleghi. Voglio sapere se siamo in presenza di un regolamento antidemocratico e antiliberale del Movimento 5 Stelle. Le chiedo se si è in presenza di un regolamento che abbia caratteristiche di tal genere e se esso possa essere compatibile con la natura democratica e liberale del Senato nel quale ciascuno di noi siede.

A me ricorda al contrario, cercando e rovistando, che quel costume e quel comportamento siano figli di un'altra Carta e di un altro articolo: non dell'articolo 21 della nostra Carta,

Quando questi principi sono in contrasto, in opposizione al documento principale, non è possibile, e quindi è vietata, la libertà di parola, di espressione. norma quella libertà essere esercitata. Reputo che i Gruppi siano diversi dai partiti e che all'interno di quest'Aula essi debbano avere regolamenti ispirati alla democrazia parlamentare alla quale siamo stati educati.

Ritengo altresì sacrosanto il diritto di ciascuno, e di un senatore in particolare, a poter esprimere il proprio pensiero con tutti i mezzi che ritiene. Ritengo altresì che l'articolo 67 della Costituzione sulla libertà di esercitare il proprio ruolo di parlamentare senza vincolo di mandato sia uno dei capisaldi della nostra democrazia e della democrazia in generale. Non ritengo però che sia possibile per quest'Assemblea entrare nelle dinamiche di un Gruppo, il quale tutt'al più ha il potere di espellere un un senatore o una senatrice e non certo quello di fargli perdere alcuna delle prerogative che, come parlamentare, ha ricevuto con l'elezione popolare, prerogative che nessun provvedimento del Gruppo potrà mai togliergli.

questo Gruppo abbia la possibilità di prendere delle decisioni, anche estreme. Il Gruppo di cui faccio parte (e neanche i partiti che hanno dato origine al Gruppo del Popolo della Libertà) non ha mai espulso nessuno, ma non possiamo sindacare su decisioni che possono essere prese da altri; possiamo solo auspicare che sia il Gruppo

io mi trovo qui a precisare esattamente cosa sia avvenuto, perché noi del Movimento 5 Stelle non abbiamo affatto leso alcun principio costituzionale. Noi alla Costituzione ci crediamo, però crediamo anche che libertà debba accompagnarsi a responsabilità. Io stesso sono qua seduto accanto alla senatrice Gambaro a dimostrazione del fatto che, qualcuno forse ipotizzava, non ci sono affatto rotture bulgare o situazioni da guerra fredda fra Corea del Nord e del Sud: c'è semplicemente il richiamo all'assunzione di responsabilità per quanto si dice e per quanto si fa. Noi tutto questo

sottoporre alla rete degli attivisti - e questo è un meccanismo di democrazia diretta e partecipata - il comportamento della senatrice, ma tutto questo nel rispetto delle libertà proprie di ogni parlamentare. Ogni parlamentare può infatti esprimere sue valutazioni, ma ciò non toglie che tali valutazioni potrebbero andare a scalfire l'unitarietà, l'omogeneità, la condivisione dei valori del Gruppo di cui è parte. Noi adesso stiamo valutando e non è stata presa alcuna decisione in merito. Ci tengo però a precisare, innanzitutto al senatore Nencini, di cui ricordo le parole quando il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha occupato quest'Aula, occupato quest'Aula, che forse sono altri i comportamenti che meriterebbero un'attenzione ancor più critica. Io mi trovo in un'Aula in cui, per esempio, degli eletti sono quasi sempre assenti

detti di suonatori di piano: dalle mie parti - e non soltanto: forse anche nel dettato costituzionale - c'è scritto che uno vale uno, quindi se è uno deve dare un voto, non due o altro; tuttavia, su questo nessuno è mai intervenuto in maniera così forte. Io sono dell'avviso che noi, con calma e certamente con pacatezza, si debba ragionare su come riscrivere le regole nel nostro stare insieme, ma le posso garantire che il Movimento 5 Stelle ha certamente a cuore le istanze di libertà di tutti quanti noi italiani eletti e innanzitutto della senatrice Adele Gambaro.

non intervengo per entrare nel merito, ma solo per dichiarare in quest'Aula il mio stupore, se così posso dire. Sarà anche previsto dal Regolamento, ma ritengo completamente irrituale e sbagliato interrompere il filo logico di una discussione che stavamo svolgendo.

Signor Presidente, non riesco (e non voglio) dimenticare che, mentre ci accingiamo a votare un atto così importante come questa Convenzione, che ha visto la sua nascita ufficiale a Istanbul, oggi in quella stessa città e in gran parte di quel Paese si vive un clima di repressione e di violenza e, come ci raccontano i *media*, in presenza di molte violenze sessuali nei confronti di giovani donne turche. La Convenzione si applica sia in tempi di pace sia in tempi di conflitto ed è una Convenzione che aspira a creare un'Europa libera...

si levi un ennesimo appello al Governo turco per interrompere la repressione ed esprimere piena solidarietà alle donne turche che hanno subito violenza e che rischiano di subirne ancora. alla Convenzione, ritengo utile sottolineare come essa sia uno strumento indispensabile per offrire una rete strutturata sia di attività che di promozione culturale, di prevenzione e di accoglienza per le donne che subiscono violenza in tutte le forme in cui essa si manifesta, così come ha ben sottolineato la senatrice Di Biasi. Sottolineo come la Convenzione delinei un percorso concreto che offre ad ogni donna la possibilità e il diritto a vivere libera dalla violenza in ogni momento e in ogni ambito della propria vita quotidiana. L'importanza della Convenzione è che non si parla di singoli progetti (di cui tra l'altro i territori italiani sono ricchi), ma si delinea un percorso che crea e struttura in modo permanente una rete di attività e di servizi, una rete costruita

non le parole, della lotta alla violenza richiede una cosa importante, che si chiama continuità delle attività e la costruzione di una rete, continuità formativa e continuità delle azioni. Serve una rete, perché sia nella prevenzione che nell'accoglienza una donna che subisce violenza ha diritto ad incontrare personale qualificato e debitamente formato, e, che incontri un vigile urbano piuttosto che un assistente sociale o un medico di pronto soccorso, ha diritto ad incontrare personale in grado di accoglierla, personale in grado di accoglierla, ma anche di orientarla rispetto ai servizi esistenti nel territorio, e personale che aiuti anche i territori a dotarsi di servizi Questa attività permanente riguarda anche la prevenzione, che va intesa come quel cambiamento necessario per il superamento degli stereotipi. In questo senso, per esempio, gli interventi nella scuola, in modo permanente, sono elementi importanti. Uscire - questo è il messaggio chiaro, il contenuto chiaro della Convenzione dai progetti per un'attività permanente e importante. In tal senso, la *task force* istituita dal Ministro è un elemento importante, e credo che anche da quest'Aula debba venire il sostegno concreto ribadendo, come hanno fatto alcuni colleghi prima di me, che anche in quest'Aula ci sono competenze importanti.

che le vittime abbiano accesso ai servizi sociali e sanitari e che tali servizi debbono disporre di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate. E allora approvare oggi la Convenzione in quest'Aula è un atto importante, ma altrettanto importante è sentirci tutti impegnati ad una coerenza e rispettare quindi un patto con le donne italiane. Occorre per esempio, anche nel decreto «del fare» e negli atti normativi che approveremo, rifinanziare le attività ed i servizi, come le case rifugio e la rete dei pronto soccorso rosa, i cui finanziamenti sono stati interrotti. Abbiamo un impegno in qualche modo, che discende naturalmente dalla Convenzione:

è in qualche modo anticipata da quello che le esperienze nei territori ormai hanno maturato da anni. Ho presente l'esperienza del mio territorio, della Provincia di Arezzo, dove ormai da più di quindici anni esistono una rete strutturata ed un lavoro permanente promosso e coordinato dalla Provincia, che coinvolge tutti i Comuni, la prefettura, le forze dell'ordine e le associazioni di volontariato. E ancora una volta, guardate, la politica nazionale e il legislatore sono indietro rispetto all'esperienza dei territori. E allora non rimaniamo ulteriormente indietro; l'impegno è di calendarizzare e di approvare rapidamente la legge sul femminicidio ed essere coerenti rispetto ai finanziamenti che necessitano per attivare questa rete e garantire i servizi necessari. Concludo dicendo che, mentre dobbiamo fare questo, dimenticarci però che quella del femminicidio è una vera e propria guerra, e questa guerra la si può vincere solo e soltanto nel cuore e nella testa delle persone. Io mi chiedo costantemente, ogni volta che penso a questo dramma, cosa succede nella testa di un uomo, quell'uomo che violenta, che perseguita, che ammazza una donna, la quale spesso è la sua donna, sua moglie o ex moglie, la sua fidanzata o la sua ex fidanzata, una donna con cui si sono condivisi sogni e intimità, con cui magari si sono generati dei figli. Un uomo che improvvisamente vede quella donna e la fa diventare quasi una sagoma di cartone contro cui sparare e contro cui infierire; cosa succede nella testa di quell'uomo? E allora io mi domando sempre più come si debba fare per portare avanti, insieme alle norme, anche quell'azione importante di promozione culturale per cui, così come diventa naturale innamorarsi, deve diventare altrettanto naturale far finire quell'amore. Si pone allora il tema di come la politica e la sua attività istituzionale e culturale debbano riportare al centro quelle parole che sono tabù, che sono appunto la sessualità e l'amore, e ridare loro dignità e spazio anche in quei luoghi in cui oggi in qualche modo è vietato parlarne, come ad esempio nelle scuole (se non è vietato, è comunque difficile). Serve promuovere una cultura dell'affettività e della sessualità non basata sul possesso, ma basata sulla libertà e sul reciproco rispetto. E la libertà non è soltanto in un ambito, ma è in tutti gli ambiti, anche - tornando al ragionamento di prima - dove si vive e si concretizza, come in Parlamento, l'attività dei Gruppi parlamentari.

penso davvero - l'ho detto anche poco fa intervenendo per altre ragioni - che questo di stasera sia un momento importante, forse addirittura uno dei più importanti, almeno nella recente storia di questa legislatura, che ci vede impegnati nella discussione per la ratifica della Convenzione di Istanbul, o meglio - io voglio chiamarla così della Convenzione per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. Anche io, come altri, credo infatti che bisogni nominare interamente il titolo della Convenzione, per darle la rilevanza che essa merita, per il significato altamente simbolico, ma anche per gli indirizzi di intervento che predispone e per le linee con le quali questo strumento fondamentale si propone di combattere e di prevenire le violenze che incessantemente si consumano sul corpo delle donne e che tuttavia non sempre

dei deputati e dei senatori della precedente legislatura (che naturalmente ringrazio), del Presidente del Senato e della presidente della Camera Boldrini, grazie al loro impegno a far sì che la ratifica della Convenzione fosse tra le prime leggi approvate dal Parlamento nel corso della XVII legislatura. Non è naturalmente irrilevante che l'Italia sia il quinto fra i 47 Paesi del Consiglio d'Europa a procedere alla ratifica della Convenzione e non è inutile ricordare - è stato già detto - che, affinché la Convenzione sia operativa, occorre la ratifica di almeno dieci Stati del Consiglio d'Europa. Questo, signor Presidente, impone al nostro Paese un onere politico e un obbligo morale: quello di farsi promotore affinché altri Stati dell'Unione europea ratifichino al più presto e nel numero più ampio possibile la Convenzione. Sarebbe questo un passo fondamentale perché la questione della violenza di genere diventi non un tema tra tanti, una postilla - pure importante - del novero più largo dei diritti della persona, ma parte integrante, costitutiva e qualificante del *corpus* di diritti umani fondamentali garantito dall'Unione alle sue cittadine. Se questo, come credo, è l'obiettivo da perseguire, si deve partire dalla constatazione che la violenza di genere va affrontata come fenomeno politico e sociale insieme; e che dunque non è soltanto il tema della prevenzione e del contrasto, peraltro fondamentale, a dover essere oggetto degli interventi legislativi dei singoli Governi europei e della stessa Unione, ma che si tratta di una questione che non può che essere affrontata alla radice e sotto più aspetti, non ultimo quello culturale. Senza questo salto di paradigma semplicemente verrebbe indebolita e revocata in dubbio la natura e la qualità della democrazia in Europa. L'Unione europea si presenta spesso più attenta ai crudi numeri degli equilibri di bilancio che ai diritti e alla loro piena attuazione, che invece si ammette vengano sacrificati alla logica del risanamento. Però si dà il caso che non sempre sia possibile che questo avvenga a costo zero per i bilanci. È in questo senso che va data piena attuazione (ed è indispensabile che il Governo fornisca assoluta garanzia circa lo stanziamento delle risorse necessarie allo scopo) alla Convenzione

comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata», com'è stato ricordato. Come si vede, è una formulazione questa, che individua con efficacia il tema della violenza di genere, ma che aiuta anche a decodificare la natura tutta politica della questione, il suo riguardare la sfera della libertà in tutti i suoi aspetti, da quelli psicologici a quelli economici, il suo essere questione appunto attinente alla sfera pubblica e a quella privata. Abbiamo tutti nella mente la vicenda terribile di Fabiana, la crudele morte inflittale da un ragazzo con solo qualche anno più di lei, che si è arrogato incredibilmente il diritto di disporre della sua vita in modo così atroce. Quale idea di sé, quale idea dell'altro da sé, del genere femminile può portare un ragazzo a ritenere di poter privare della vita una donna come fosse cosa sua e di nessuna importanza? Finalmente negli ultimi anni ci si è resi conto che gli omicidi come quelli di Fabiana non sono solo tragedie personali, ed è diventato appunto di uso comune il termine «femminicidio». Ecco, in questo sostantivo c'è il nocciolo della questione. Che dietro le violenze di genere, fino alla forma estrema del femminicidio, ci sia la drammatica questione del mancato riconoscimento dell'altro da sé che è il genere femminile e che dunque il lavoro da fare sia tanto enorme quanto indilazionabile e che riguardi moltissimo la sfera culturale,

Ma proprio in questa direzione sono fondamentali gli interventi che la Convenzione raccomanda sul terreno della prevenzione. È da lì, dai primi anni del percorso formativo che si può innestare un'educazione civile che contrasti i tanti danni che la reificazione del corpo femminile a scopi commerciali e pubblicitari oppure uno stereotipo di subalternità del genere femminile, che - non dimentichiamolo - è ancora profondamente radicato nel senso comune maschile, hanno prodotto. Tuttavia, occorre ricordare come spesso la condizione materiale ed anche la concreta socialità delle donne a condizionare e a determinare percorsi, destini e scelte, come cioè la possibilità di sottrarsi a violenze e abusi sia direttamente proporzionale all'indipendenza e all'autodeterminazione delle donne. Che possibilità avevano - lasciatemelo chiedere così le cinque donne che nell'ottobre del 2011 sono morte a Brindisi, sepolte dal crollo dello scantinato in cui lavoravano per meno di quattro euro l'ora? Che possibilità aveva la più giovane di loro, che aveva soltanto 14 anni? Voglio ricordarne in quest'Aula il nome: si chiamava Maria Cinquepalmi. Certo non è morta direttamente di violenza maschile, ma non è morta forse di necessità, di solitudine sociale, della impossibilità di scegliere che fare della propria vita? Insomma, che alla radice della violenza vi sia una drammatica disparità, un'asimmetria intollerabile che attiene all'ordine sociale, che riguarda anche e soprattutto la minaccia che la libertà e l'autonomia femminile possono portare, secondo il punto di vista maschile, ad un ordine simbolico consolidato che non ammette altro da sé, mi pare un fatto indiscutibile. Ma del dato che la violenza di genere copre anche ingiustizie, sfruttamento, esclusione di cui le donne sono fatte segno perché più esposte, più ricattabili, più sole, dovremmo, anche attraverso lo strumento della Convenzione, trarre occasione di riflessione. In questo senso, dobbiamo guardare con sgomento ai dati dell'occupazione femminile, soprattutto di quelli meridionali. Al Sud lavora una giovane donna su quattro. La SVIMEZ, in un suo studio recente, ha descritto come, anche per effetto del marcato processo di distruzione del tessuto produttivo indotto dalla lunga crisi economica, le giovani donne meridionali che sono ormai mediamente più scolarizzate delle coetanee del resto del Paese - non abbiano altra scelta se non l'emigrazione o la regressione forzata, per mancanza di lavoro, ad un ruolo di casalinghe che apparteneva alle loro nonne ed era stato superato dalle loro stesse madri. Che questo si configuri come una gigantesca regressione civile per il Paese e una perdita intollerabile per la società italiana mi pare fin troppo evidente per doverlo sottolineare con altre parole. Insomma, il fatto che il tema della violenza di genere, della mancanza di autonomia, della subalternità delle donne vada affrontato con un complesso di strumenti è argomento che la Convezione mette a tema offrendo ai Governi una griglia operativa e una direzione di marcia; tuttavia spetta alle nostre scelte politiche non solo compiere un'operazione simbolica, ma costruire concretamente le condizioni per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che costituiscono le condizioni dentro cui matura la violenza di genere contro le donne. Anche per questo una misura come il reddito minimo incondizionato restituirebbe alle donne - anche alle donne - la possibilità di sottrarsi alla subalternità, ai ricatti e ai soprusi a cui ho fatto riferimento. onorevoli senatori e senatrici, è intollerabile che sia stata cancellata nella scorsa legislatura la legge sulle dimissioni in bianco che dava la possibilità di tutelare l'autodeterminazione della donna, la sua possibilità di scegliere tra maternità libera e consapevole e la possibilità di avere insieme un lavoro e un ruolo sociale. Allora, mi chiedo con voi; ha senso ratificare la Convenzione di Istanbul e non reintrodurre quella legge? Allo stesso modo è necessario garantire che le donne possano usufruire di un irrinunciabile presidio come la legge n. 194 del 1978 e insieme di tutte quelle tutele sociali che invece vengono colpite per prime ad ogni manovra di bilancio da molti anni a questa parte, e in misura tale che soprattutto al Sud il *welfare* è di fatto azzerato, con effetti deleteri soprattutto sui presidi di frontiera come gli sportelli antiviolenza. antiviolenza. Signora Presidente, riteniamo che da qui si debba partire: oggi con la ratifica della Convenzione di Istanbul, domani continuando a perseguire con determinazione la strada che libera le donne dall'ipoteca di una libertà diseguale e la nostra società dalla piaga della violenza di genere.

Troppo spesso nel nostro Paese si manifesta una nuova moda, una moda secondo la quale i processi vengono fatti, prima in televisione, poi nelle aule di giustizia. Purtroppo è una moda in continua crescita. Io per cultura non ho mai amato né i processi sommari né i processi di piazza, e tanto meno mi entusiasmano quelli televisivi, anche perché in questa nuova moda spesso pescano a piene mani i mezzi di informazione, e in un clima simile va da sé che tutte le garanzie costituzionali del giusto processo diventino delle variabili indipendenti. Di questo sistema perverso credevo di aver visto tutto, invece è accaduto qualcosa di nuovo. Giovedì 6 giugno 2013 Michele Santoro presenta una puntata speciale di «Servizio Pubblico Più» dedicata a un fatto molto grave e importante per il nostro Paese: la trattativa Stato-mafia. Non un processo di cinque, dieci o vent'anni fa, ma un processo in corso e appena iniziato. Chi partecipa a quella trasmissione, signora Presidente? Evito di ricordarle i nomi dei professionisti dell'antimafia, quelli che sono in SPE (per chi non conosce l'acronimo militare: in servizio permanente effettivo). A quella trasmissione partecipa un magistrato (anzi, sono due), e non è un magistrato fuori corso: guarda caso, è proprio il che esercita e regge l'accusa nel processo sulla trattativa Stato-mafia, Antonino Di Matteo. Lui - proprio lui! parla del processo sulla trattativa Stato-mafia e di fatti riguardanti altro processo, la cui sentenza è attesa per il prossimo mese di luglio, quello che riguarda il generale Mori, strettamente legato al processo sulla trattativa Stato-mafia. Se lei solo per un istante pensasse che questo fosse tutto, andrebbe ancora una volta delusa, perché a quel processo partecipa un altro magistrato (intendo il processo televisivo: quando la *fiction* supera la realtà), la realtà), ossia il dottor Piergiorgio Morosini. Allora, se stiamo nella *fiction*, possiamo immaginare che il pubblico ministero, essendo parte del processo, potrebbe avere un diritto quasi di cittadinanza, ma se parliamo del dottor Piergiorgio Morosini, parliamo del giudice terzo, di quello che dovrebbe garantire lo Stato, lo Stato Concludo subito, signora Presidente. Attraverso la funzione che lei svolge, vorrei che questa mia interrogazione potesse rivestire quel carattere di urgenza che questi fatti meritano.

oggi, in questo momento, voglio ricordare l'ennesima donna uccisa dalla barbarie. Questa volta purtroppo è capitato anche alla mia provincia (dico "anche" perché il problema è trasversale e sappiamo tutti che attraversa ogni strato sociale e ogni comunità geografica). È accaduto qualche giorno fa in un luogo sacro, in un posto in cui ci si sente sicuri: a scuola, dove mandiamo i nostri figli, dove gli insegnanti e tutto il personale vanno a lavorare serenamente;

ma occorrono due cose fondamentali. Una cosa molto prosaica, che sono i soldi perché, come si dice a casa mia, «senza soldi non si canta messa». Purtroppo, è stato detto e ribadito, che sono pochissimi i centri di accoglienza, i centri di ascolto e le case di protezione per le donne. Vi assicuro che in Sicilia ce ne sono ancora meno.

Possiamo soltanto adoperare queste figure generose che possono avere, a volte, la professionalità, ma non sempre il tempo, e ricordo che sono necessari tempi stabili e sicuri e professionalità altrettanto certe. Pongo quindi alla vostra attenzione il problema. In questi giorni

perché se le donne stanno meglio, è la comunità che sta meglio. Le donne che subiscono violenza, infatti, o si ammalano, e hanno bisogno di farmaci ed interventi, o muoiono e ci sono i figli che subiscono e crescono con il dramma della violenza assistita. L'intervento di prevenzione è perciò assolutamente necessario e non può essere più a macchia di leopardo, ma deve essere diffuso in tutto il Paese. Non è possibile che il Paese venga diviso ancora una volta anche per questo dolore in un Paese di serie A e in un Paese Abbiamo tutti diritto ad avere lo stesso tipo di assistenza. Ma questo non basta. Questa era una prima riflessione. La seconda riflessione è culturale. È stato detto e ribadito che non basta un decreto, non basta una norma e non bastano i centri.

una giornata di riflessione. Annuncio in questa occasione che sto presentando un disegno di legge volto a prevedere una giornata durante l'anno scolastico, forse nel mese di ottobre (poi deciderà chi deve decidere),

Signora Presidente, distinti colleghi, il 22 maggio, citando Matteo Iori, presidente dell'associazione CONAGGA, posi alla vostra attenzione il conflitto di interessi tra politica e industria del gioco d'azzardo e il trasparire di una precisa volontà politica di assegnare nuovamente la delega al sottosegretario del PdL Alberto Giorgetti. Così dissi e così è avvenuto: non solo ha avuto la delega al gioco d'azzardo, ma anche un più ampio potere sulle questioni di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, da cui l'erario emunge annualmente decine di miliardi ambita, pregiata, dunque. Ma quali sono i suoi meriti? Essere gradito all'industria del settore? Come dice Iori, Giorgetti gestì la delega per i giochi durante l'ultimo Governo Berlusconi e fu particolarmente apprezzato dalle industrie del gioco per la sua capacità di aiutare nell'introduzione di tanti nuovi giochi d'azzardo: la *videolottery*, il *win for life*, i concorsi aggiuntivi del superenalotto, il bingo a distanza, il *poker on line* in solitario e molti altri. Il volume di giocate ebbe una impennata, con un incremento del 30 per cento in un solo anno, dal 2010 al 2011. Ricordo che a livello epidemiologico la diffusione, la disponibilità e la facile accessibilità ai punti di gioco sono fattori che aumentano la dipendenza patologica. Secondo stime restrittive, i giocatori patologici sono 700.000 almeno e vivono in famiglie dove tutti soffrono, anche i bambini. Da uno studio del Dipartimento politiche antidroga, poi, emerge che quasi l'8 per cento dei ragazzi quindicenni gioca verosimilmente in modo problematico. Ciò dimostra come siano illusori i controlli attuali e quale epidemia ci dobbiamo preparare ad affrontare. Di questo *business* allo Stato arrivano 8‑10 miliardi l'anno, ma il gioco d'azzardo sottrae risorse ai consumi di generi alimentari e di beni primari: l'economia langue e le imprese muoiono. Anche l'erario perde, con il mancato introito di Uno studio dell'università di Neuchâtel stima in oltre 6 miliardi i danni sociali e sanitari causati dal gioco d'azzardo. Perché dunque perseguire questa assurda espansione? Fondazioni e associazioni *non profit* hanno implorato di invertire la rotta e che la delega non andasse a chi aveva spinto alla diffusione di questi cosiddetti giochi, invece proprio Giorgetti è stato scelto dal Governo Letta. Per quale motivo, nonostante le autorevoli proteste? Come si intende sgomberare il campo dai dubbi di conflitto di interesse che hanno investito diversi esponenti del Governo? domande alle quali i Ministri dovranno ora rispondere: un'interrogazione verrà presentata a breve.

Signora Presidente, vogliamo denunciare un fatto molto grave. Stiamo assistendo in questi giorni a una tragedia immane, un'emergenza umanitaria che coinvolge donne e bambini. Nel mar Mediterraneo, migliaia di persone mettono a rischio la vita nel nome di una speranza che difficilmente sarà raggiungibile. La situazione è gravissima e il nostro Paese non può farsi carico ancora una volta da solo, in maniera unilaterale, del problema. Dobbiamo chiedere immediatamente l'intervento dell'Unione europea. L'Unione europea ha le mani sporche di sangue, altro che Nobel della pace! che l'Unione europea la smetta di girare la testa da un'altra parte, è ora che l'Unione europea onori gli impegni presi con il nostro Paese. Chiediamo a lei che si faccia portavoce presso il Governo affinché venga a riferire subito in Aula su questa situazione. *(Applausi del ci permettiamo di dare un consiglio. Un Ministro dell'interno, del quale non faccio il nome, in un recente passato, ha messo in campo un piano straordinario che di fatto bloccava gli sbarchi. Un piano straordinario da molti criticato

quel piano straordinario per lo meno garantiva quello che oggi l'Unione europea non riesce a garantire: la carità cristiana. in questi giorni 6.000 metri quadrati di mais OGM sono stati seminati a Vivaro, in Friuli. Ben due procure, Padova e Pordenone, si erano già espresse negativamente a proposito di un agricoltore che qualche anno fa aveva seminato mais OGM. Anche la Corte di cassazione nel marzo del 2012 ha ravvisato nella condotta di chi semina mais OGM l'integrazione di un reato. La vicenda OGM va avanti ormai da troppo tempo e questa deve essere l'occasione per chiudere definitivamente una questione sulla quale cittadini e agricoltori, rappresentanze economiche e sociali, Regioni e Parlamento si sono espressi già tantissime volte. Ricordo anche che la messa a coltura di OGM costituisce un'attività pericolosa, come da codice dell'ambiente, e prevede azioni di prevenzione del danno ambientale. Alla luce e nel rispetto delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 settembre 2012 e del 18 maggio 2013, il diritto di coltivare organismi geneticamente modificati deve convivere con il diritto dello Stato di condizionare la coltivazione ad adeguate misure di coesistenza con l'agricoltura tradizionale o biologica, al fine di evitare ogni possibile contaminazione di tali produzioni e conseguenti danni economici. La legittimità della messa a dimora di OGM continua ad essere subordinata alla verifica che le concrete condizioni di tale coltivazione siano idonee ad evitare la contaminazione con altre produzioni. Chiediamo, come Movimento 5 Stelle, al Governo il completamento della procedura di adozione della clausola di salvaguardia, come peraltro già sollecitato da tutti i Gruppi parlamentari al Senato con una mozione votata all'unanimità e come già fatto da tempo in diversi Paesi. In particolare, chiediamo al Ministero dell'ambiente di emettere un'ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell'agroecosistema, in forza dell'articolo 8 della legge istitutiva dello stesso Ministero.